aveva dato l'opportunità, l'onere e l'onore ai parlamentari di contribuire al recepimento delle direttive europee e di commentare l'adozione dei regolamenti.

la normativa europea ormai costituisce il 70 per cento delle nuove leggi e sappiamo bene come queste spesso cozzino con gli interessi del nostro Paese. È uno strumento importante per dare l'opportunità ai parlamentari - soprattutto

modifica erano solo una buffonata, perché sapevamo già dall'inizio che nulla sarebbe stato accettato e che nessun emendamento sarebbe stato accolto semplicemente perché non si vuole ripassare all'altra Camera. Stigmatizzo pertanto questo comportamento assolutamente privo di senso; fa perdere tempo alle Commissioni

Alla Camera avevamo proposto talune modifiche perché sapevamo già che qui nulla sarebbe potuto essere accolto; in particolare, avevamo chiesto di togliere il monopolio alla SIAE per quanto riguarda la direttiva sui diritti d'autore. Sappiamo che, purtroppo, in Italia, vige questo monopolio. Alla Camera avevamo presentato

in questo momento mi rivolgo specialmente al relatore, affinché ponga una particolare attenzione su questa direttiva. Abbiamo parlato della direttiva sull'etichettatura. Nel testo della legge europea eravamo riusciti a fare ritirare al Governo il famoso articolo 3, che impediva di indicare in etichetta l'origine della materia prima. Eravamo contenti, abbiamo fatto comunicati stampa, eravamo tutti felici e invece avete reintrodotto la norma con il disegno di legge di delegazione europea, quindi avete nuovamente svenduto le nostre eccellenze alle multinazionali. Mi rivolgo a chi ieri ha fatto presente che noi italiani abbiamo aziende di trasformazione molto importanti.

potrà così scegliere se consumare un prosciutto di Parma con le cosce che provengono dalla Polonia oppure uno nostrano. Si tratta semplicemente di tutelare la filiera e di dare libertà

le eccellenze agroalimentari e invece di andare in infrazione per quanto riguarda la gestione virtuosa dei rifiuti è un'infamità: è un'infamia anche per i vostri cittadini. Noi preferiamo andare in infrazione per tutelare l'agroalimentare e vogliamo invece che risolviate le infrazioni per quanto

legge n. 2345** Onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno riguarda l'approvazione della legge di delegazione europea 2015, europea 2015, che contiene più di una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Si tratta quindi di un provvedimento, che, con cadenza annuale, adegua il nostro ordinamento alle norme prodotte dal legislatore europeo, in questo modo l'Italia ottempera agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea. Di fatto il Parlamento italiano si ritrova a recepire e dare attuazione agli atti europei in maniera del tutto passiva, e, talvolta, per non dire troppo spesso, la pura e semplice immissione delle regole europee nel nostro ordinamento, va ad se non accettare pedissequamente le proposte dell'Unione europea. Questo va a incidere in maniera negativa nei settori cruciali della nostra economia e della nostra società. Noi siamo critici - molto critici - nei confronti di questa prassi legislativa, del tutto incurante delle peculiarità e specificità del nostro sistema Paese. Vi sono altresì dei gravi profili critici all'interno del disegno di legge

il nostro *made in Italy*: abbiamo svenduto la nostra qualità, la nostra etichetta e le nostre peculiarità. Stiamo vivendo un momento storico negativo e mi auguro che gli agricoltori a suo tempo sapranno capire che questo Governo

in materia di etichettatura. Si legge che il recepimento può comportare anche l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali: complimenti!

in quanto non dovremmo in alcun modo cancellare i riferimenti normativi interni che rappresentano gli unici strumenti per difendere e sostenere l'eccezionalità del *made in Italy.* Italy.* Piuttosto, dovremmo fare in modo che le istituzioni europee e gli Stati membri si adeguino alla normativa italiana in materia. Per quanto riguarda l'obbligo di indicare sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, negando la possibilità di indicare invece il luogo di produzione,

Se oggi il vino vanta delle caratteristiche e riusciamo a venderlo come un prodotto di grande qualità - il migliore al mondo - è grazie a queste etichette che ne hanno garantito l'origine, la produzione, il luogo

un danno enorme. Altri punti, che ho già citato e che ho riscontrato nella legge europea, riguardano anche il fatto che si individuano come organi di vigilanza la Banca d'Italia e la Consob. In questo senso, a mio avviso si sta facendo un altro grande errore, perché abbiamo visto che le attività di controllo a cui sono preposte non sono state condotte con adeguata efficacia comunque, il loro risultato è stato alquanto discutibile. Abbiamo visto come, nelle fattispecie introdotte, si conferisce alla Banca d'Italia questa facoltà e questa possibilità quando

Proprio per questo, se importiamo prodotti, dobbiamo essere certi della differenza tra il nostro prodotto, italiano, garantito, e un prodotto che viene dall'estero. Dovremmo preoccuparci ancora di più di questo. Pare però che non si capisca l'importanza di indicare nelle etichette il luogo di produzione. Per assurdo, potremmo anche accettare che il confezionamento avvenisse in un altro Paese, a sapere qual è il luogo di produzione che ne determina la qualità, le peculiarità e le caratteristiche che prima ho citato. Ma questo sembra non essere capito, o forse davvero c'è un atteggiamento di sudditanza verso questa Europa che nulla sta dando al nostro Paese.

che incidono, se solo li dividessimo per il grano tenero, per 10 centesimi al quintale? Non oso suddividerli per il mais, per l'orzo, per il grano duro, altrimenti parleremmo solo di due o di due o tre centesimi per quintale. Ma pensate che siano messi così male gli agricoltori italiani da aver bisogno dell'elemosina che proponete loro con questo piano cerealicolo da due o tre centesimi per quintale? No, signori vi sbagliate. Gli agricoltori italiani, se ancora oggi praticano l'agricoltura, è perché hanno tanta dignità. Ma sono stanchi. Sono stanchi di essere trattati in questo modo da un Governo che non sa capire i veri problemi dell'agricoltura e da un Ministro che non si presenta neanche in Aula quando si parla di leggi

sono stati messi nella rete, sono caduti nella rete di questo Governo. Però vi sbagliate se pensate di risolvere i problemi dell'agricoltura in questo modo perché gli agricoltori sono, innanzitutto, delle brave persone che hanno nella famiglia

anche il Governo e il presidente della Commissione 14a Vannino Chiti, che ha sempre governato questa Commissione con grande equilibrio e cui tutti noi siamo riconoscenti per come si è mosso anche in occasione di questo percorso della legge di delegazione.

che ci faceva pensare all'Europa come alla panacea per tutti i mali, ma che dimostrava nei fatti concreti una certa superficialità. Questo ha condotto ad alcune scelte che oggi scontiamo. Oggi ci troviamo a dover risalire la corrente per errori fatti per un eccesso di faciloneria nell'approccio ai temi europei e però ci troviamo in una condizione per certi aspetti opposta: un euro-scetticismo ipercritico e, a sua volta, superficiale. Oggi l'Europa viene spesso utilizzata per polemiche di bassissima lega a scopi interni, che non tengono conto della realtà economica, sociale e imprenditoriale, né dell'Unione europea, né del nostro Paese. Sia l'europeismo acritico che l'euroscetticismo ipercritico mi sembrano due espressioni provinciali del nostro Paese,

protagonisti attivi, o coloro che fanno in prima persona la politica europea e non quelli che devono semplicemente averne il riflesso più o meno indiretto. Non abbiamo nulla da chiedere, né da mendicare. Chiediamo soltanto il rispetto dei Trattati che abbiamo liberamente sottoscritto e una loro applicazione lungimirante volta a rafforzare l'Unione e non a indebolirla. C'è stato molto strabismo nella lettura dei Trattati che ha portato a vedere solo l'aspetto della stabilità, anziché anche quello della crescita. C'è un merito che va riconosciuto al Governo Renzi: ha saputo imporre ai nostri *partner* e interlocutori europei una visione più equilibrata e sana, tanto più necessaria in una fase come quella che abbiamo vissuto che è stata caratterizzata e connotata da una lunga fase di recessione dovuta alla crisi finanziaria. Per fare questo e riuscire ad ottenere il riequilibrio del tema della stabilità e della crescita è stato necessario recuperare la credibilità, che ‑ mi spiace dirlo ‑ il nostro Paese aveva perso sia per la sua incapacità di mantenere gli impegni assunti, *in primis* nella riduzione del debito pubblico, sia per i comportamenti eccentrici di alcuni nostri rappresentanti e per il discredito personale che si rifletteva, a causa loro, sull'intero Paese. Si tratta di un discredito che, a volte, temo potrebbe ritrovare fiato, sentendo i toni sguaiati di alcune opposizioni, che abbiamo ascoltato anche oggi in Aula e che non fanno bene né alla serietà del dibattito, né all'immagine dell'Italia. Oggi l'Italia ha recuperato totalmente la propria credibilità sul piano personale dei propri rappresentanti, grazie all'opera del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti del suo Governo. Lo abbiamo visto all'indomani della si è riunito a Berlino un trio composto da François Hollande, da Angela Merkel e da Matteo Renzi. Non avevamo mai visto, in passato, Presidenti del Consiglio italiani chiamati in una fase di crisi acuta, come quella che si è verificata dopo la Brexit. Lo abbiamo visto anche nella capacità di proporre un nuovo rilancio dell'Unione europea, che troverà un punto di forza nell'incontro di Ventotene di fine agosto, e lo vediamo anche nella proposta di celebrare e rilanciare l'Unione europea in occasione del settantesimo anniversario dei Trattati, a Roma, nel marzo del 2017. Stiamo facendo molto per recuperare, anche sul piano dell' attendibilità degli impegni assunti di questo è stato dato atto da parte della Commissione europea. Vorrei ricordare che, pochi giorni, fa la Commissione europea ha ringraziato l'Italia, evidenziando che c'è stata una riduzione, dalle 119 procedure di infrazione che erano aperte nei confronti del nostro Paese nel marzo 2014 - ovvero nel momento in cui

del 34 per cento, che la Commissione stessa ha detto essere senza precedenti. L'Italia oggi ha fatto registrare le migliori *performance* in assoluto, rispetto a qualsiasi altro Paese europeo. Bene anche l'utilizzo dei fondi strutturali, che, nonostante un avvio francamente disastroso, oggi sono stati totalmente utilizzati e rendicontati. Anche questo è un grande merito del nostro Governo, che ci fa recuperare in credibilità. È questa anche la ragione per la quale è importante approvare in tempi rapidi esame ed è importante che si sia realizzata questa collaborazione tra noi e la Camera dei deputati, per consentire non soltanto l'approvazione del provvedimento, ma anche la presentazione di una nuova legge di delegazione, nel secondo semestre dell'anno.

avviare un regionalismo flessibile, nel quale le spese pazze di alcune Regioni - che raggiungono un debito pubblico regionale del 200 per cento e, in un caso, anche del 300 - indeboliscono fortemente la capacità di operare del nostro Governo, nella fase di contenimento del debito pubblico, che è il principale peccato che ci viene rimproverato. Con l'approvazione della riforma in autunno da parte del popolo italiano, sulla quale non abbiamo dubbio alcuno, saremo in grado di portare un ulteriore tassello di forza nella nostra politica e di far valere maggiormente gli interessi del nostro Paese. Così come noi ci impegniamo a rispettare le regole, anche gli altri Paesi devono fare lo stesso. La Germania deve aumentare gli investimenti e ridurre il *surplus* commerciale: tale sfasatura rende infatti il motore europeo completamente sfasato e di La Francia deve rispettare il rapporto tra *deficit* e PIL, che da anni non viene rispettato ed è fuori controllo. Bene la clemenza della Commissione europea, che ha proposto ieri, nei confronti di Spagna e Portogallo, di tollerare un provvisorio sforamento dei parametri di Maastricht, in considerazione dei grandi sforzi e delle riforme strutturali importanti che sono state approvate. È un bene anche che la Commissione abbia intimato alla Polonia di correggere il suo sistema di garanzie costituzionali entro tre mesi: infatti l'accento sul fatto che i Trattati europei devono essere rispettati non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo dei valori nei quali ci riconosciamo. Il fatto che ci siano oggi dei Paesi che pongono dei problemi gravi dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e delle garanzie, anche nei confronti degli immigrati, è un punto su cui l'Unione europea non può più chiudere gli occhi e abbozzare. Noi pensiamo che chi non rispetta i principi europei, tutti i principi europei, debba vedersi sospesi i benefici, a cominciare dall'assegnazione dei fondi strutturali. Noi siamo una comunità che deve condividere le responsabilità e i benefici, ma chi non condivide le responsabilità non può condividere nemmeno i benefici: questo è un punto che va affermato e che darà dignità e forza alla battaglia politica che l'Unione europea sta portando avanti. signor Presidente, per quanto riguarda il tema di cui oggi si parla molto, il tema della Brexit, è importante che il Regno Unito avvii al più presto la procedura di attuazione dell'articolo 50, perché, in questa fase di incertezza e instabilità che caratterizza la storia europea, questo percorso non non è positivo e crea ulteriori turbolenze ed ulteriori dubbi per il futuro. Io credo che dalla vicenda della Brexit sia possibile, per l'Unione europea, recuperare delle occasioni importanti. Ci sarà una maggiore coesione la zona euro verrà a coincidere maggiormente con l'Unione europea; da qui potremo trovare una maggior coesione anche sulle politiche economiche. io credo che oggi, anche grazie al dibattito che c'è stato in quest'Aula, grazie agli interventi mi sembra cristallini e chiarificatori su certe polemiche del tutto strumentali (l'abbiamo sentito anche dai toni), contributi del senatore Dalla Tor, della senatrice Bertuzzi, della senatrice Pignedoli e del senatore Mancuso, che hanno messo a tacere questo modo strumentale di utilizzare la politica europea per finalità strettamente elettorali interne ed hanno ben chiarito il senso della legge della legge di delegazione sull'articolo 5, stiamo rendendo un servizio importante sia al nostro Paese sia all'Unione europea. Noi vogliamo stare a testa alta nell'Unione europea, vogliamo far rispettare i principi e i Trattati, così come li vogliamo rispettare noi,

Signor Presidente, colleghe e colleghi, ricordo preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012 che, nel modificare l'articolo 81 della Costituzione e nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste, appunto, «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 15, comma 10, della medesima devo altresì segnalare che il testo iniziale della proposta, di iniziativa parlamentare, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, per cui è necessario darne conto, sia pure per sommi capi, atteso l'elevato numero di modifiche sia dei contenuti della proposta iniziale che delle numerose innovazioni successive, peraltro approvate nello spazio di pochi giorni. Insieme alla integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale, la proposta provvede al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare, viene posposto al 27 settembre (al 30 settembre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione bilancio della Camera), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio, disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento, che non prevede al momento

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta in sede referente (lettera *c-bis)* del comma 5), che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. La *ratio* dell'intervento è di tutta evidenza. Sui contenuti del DEF si interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nei testo iniziale ma notevolmente modificati durante l'esame in Commissione alla Camera, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al benessere equo e sostenibile. In particolare si dispone che, in apposito allegato al DEF, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. A tal fine, il successivo articolo 14 istituisce un apposito comitato presso l'ISTAT. Si prevede inoltre (comma 10-*ter*) che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità, ma nell'articolo 1 della proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità «di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento». Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera si è specificato che i *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei documenti di bilancio siano in formato aperto e riutilizzabile ai sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale. L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito - com'è noto - dalla nuova legge di bilancio che, nell'articolo 2, viene articolata in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni da introdurre secondo le condizioni e i limiti esposti nella proposta di legge. Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame va ricordato anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggiore elasticità gestionale, spesso introdotta da alcune norme in via transitoria. In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti che qui non si dettagliano, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sia stato anche oggetto di un ulteriore arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2 in commento) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto dalla legge di contabilità (articolo 38-*septies*) a opera di uno dei due recenti decreti legislativi (il L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi e ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni, l'esame condotto in Commissione alla Camera è stato particolarmente incisivo, e ha portato a un significativo miglioramento del testo iniziale. delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si contemplava, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscano diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsi l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi. Con riferimento alle leggi di spesa, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri, si esclude che si possa ricorrere all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene in corso di esercizio decurtato ai sensi di disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Parimenti è stato confermato l'analogo divieto disposto dalla proposta di legge anche per la quota del cinque per mille del gettito IRPEF, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Tralasciando gli articoli 4 e 5, importanti novità sono state decise nel corso dell'esame in prima lettura, anche in merito agli aggiornamenti degli istituti contabili e ai profili gestionali propri del bilancio e della contabilità generale dello Stato, nonché alle modalità di redazione dei documenti conoscitivi, con l'inserimento degli articoli da 6 a 15. Con l'inserimento dell'articolo 6, in particolare, sono state apportate importanti modificazioni e integrazioni alla disciplina degli impegni contenuta nell'articolo 34 della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 2 del recente decreto legislativo n. 93 del 2016, assicurando adeguata pubblicità "periodica" alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento. L'articolo 8, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 44 («Definizione dei saldi di cassa») della legge, laddove la norma vigente prevede l'emanazione di un decreto *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze per predefinire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi, in coerenza con principi e regole prefissati a livello internazionale. L'aggiunta approvata poi con l'inserimento dell'articolo 44-*quater* alla legge di contabilità, disposta con l'articolo 9, ha consentito di definire una rigorosa procedura ai fini dell'autorizzazione all'apertura di gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni statali, allorché le stesse siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale, e dunque al di fuori del circuito di tesoreria erariale. Infine, il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame della Camera, con l'inserimento dell'articolo 15, reca il posticipo di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2, della legge n. 196 del 2009, già più volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest'anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi nn. 90 e 93 già citati, che compongono nel loro insieme un *corpus* normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016. In questo modo verrà ricondotta a un unico testo l'intera disciplina vigente in materia di contabilità Ho terminato e non manco di ricordare che, per ulteriori profili di interesse, si fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio, che ringrazio Grazie

necessita di ben poche aggiunte. L'analisi del lavoro svolto da Camera e Senato su questo importante tassello - l'ultimo che ci accingiamo a votare e che è parte di un complesso mosaico che raffigura un nuovo assetto della contabilità pubblica - è quanto mai esaustiva e importante. L'insieme delle nuove regole, sia per la redazione dei bilanci di istituzioni ed enti, sia per le scelte pubbliche sulla programmazione economica e sul reperimento e l'allocazione delle risorse finanziarie, si inserisce in tutta questa importante riflessione e approfondimento, nonché nella capacità del Parlamento di riformare lo strumento più importante dell'azione politica di qualsiasi Governo. un nuovo assetto contabile che si è venuto strutturando per un insieme intricato di questioni, alcune esogene e altre endogene alla precedente disciplina contabile; non solo, quindi, per la necessità di definire una nuova *governance* economica europea, iniziata con l'individuazione del cosiddetto semestre europeo, con i vari *compact* e, per noi, con la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio (anche se si tratta più precisamente di un equilibrio), e per dare una risposta ferma, condivisa e a suo tempo immediata alla crisi che dal 2008 ha investito la finanza pubblica continentale. è anche l'esigenza di rivedere e riordinare la previgente disciplina contabile, frutto di una stagione iniziata con la prima grande riforma del 1978 e proseguita con alcune modifiche, peraltro molto significative, che si sono susseguite nel corso di quasi un trentennio; una una stagione terminata con la ormai lontana legge n. 196 del 2009, che però già conteneva i prodromi di quella revisione, di quel riordino che è alla nostra attenzione da qualche anno. alla legge cosiddetta rinforzata del 2012 di attuazione del pareggio di bilancio, all'attenzione del Parlamento, si sono susseguiti più recentemente diversi provvedimenti previsti dalla legge di contabilità e dalla legge rinforzata

necessitano di una certa durata, un po' come quelle della Costituzione, e soffrono i cambiamenti repentini - dando luogo a un risultato sostanzialmente condivisibile, pur non mancando ragioni per esprimere qualche riserva di una certa rilevanza. Penso - ad esempio - al provvedimento che ha introdotto l'impegno delle pubbliche amministrazioni a perseguire l'equilibrio dei bilanci. È scontata la necessità di semplificare ed efficientare, anche per sostenere gli investimenti, la gestione degli enti territoriali, segnata dal Patto di stabilità interno e da complesse regole contabili. Tuttavia, perseguire l'equilibrio di bilancio attraverso un unico saldo finale tra entrate e uscite, sopprimendo il vincolo, attualmente invece ancora previsto, del pareggio di parte corrente, mi sembra una scelta incauta, in quanto la sua eliminazione comporta l'indebolimento delle garanzie per il corretto raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; una preoccupazione peraltro condivisa da più parti, anche dalla Corte dei conti. È da tempo, ormai, che nelle sedi più disparate (istituzionali, accademiche, professionali) è emersa la necessità di rivedere, nella logica e nei contenuti, l'attuale sistema che annualmente porta alla programmazione finanziaria e alla decisione di bilancio. Grazie allo spirito di positiva collaborazione che ne ha segnato l'*iter* alla Camera - collaborazione che si è riproposta in Commissione qui al Senato, nonostante l'esigenza di una sua rapida approvazione questo provvedimento contiene alcuni elementi per me certamente rilevanti, a cui hanno contribuito, come sempre in modo puntuale, i Servizi studi del Senato e il lavoro tecnico svolto in Commissione bilancio. per così dire, di scenario, è l'ulteriore passo in avanti compiuto per ridurre sempre più la rigida struttura amministrativa del bilancio, più flessibile, più adeguata alle esigenze dell'azione pubblica, del decisore pubblico, investito dell'onere di decidere sul quanto e sul come utilizzare le risorse pubbliche a disposizione. Legato a questo aspetto, mi sembra rilevante il superamento della natura formale della legge di bilancio. Negli anni passati abbiamo spesso sottolineato le difficoltà e le ricadute negative di una decisione di bilancio imperniata su due diversi documenti. Oggi l'unificazione della legge di bilancio e quella di stabilità, resa possibile dal venir meno del carattere formale del bilancio stabilito dal soppresso comma 3 dell'articolo 81 della Costituzione, consente di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come avviene attualmente. Oltre alla maggiore compiutezza del ciclo di bilancio, altro aspetto che ritengo significativo è la maggiore attenzione alla informazione, sia quella collegata ai contenuti dei documenti, come ad esempio il dettaglio sull'andamento dei settori di spesa previsto nel DEF, sia quella collegata ai nuovi strumenti conoscitivi a disposizione del Parlamento. Correlato al tema della trasparenza è l'eliminazione delle clausole di salvaguardia, che ritengo molto positiva. Ho sempre messo in evidenza l'assurdità di un meccanismo che prevede l'aumento automatico di imposte e tasse a copertura di oneri eccedenti le previsioni, sono soddisfatta della procedura che investe anche le Camere nel reperimento di risorse ulteriori. Certo, anche questo provvedimento non è immune da critiche. Per conto nostro, abbiamo voluto sottolineare due punti che dovrebbero essere considerati in maniera meno frettolosa, e lo abbiamo fatto con due emendamenti. Il primo, in materia di copertura delle leggi di spesa, è volto a sopprimere la norma che prevede la possibilità di modificare parametri che determinano l'evoluzione di alcune tipologie di spesa, ampliando così le attuali modalità attraverso le quali fornire copertura finanziaria ai nuovi o maggiori oneri recati da disposizioni legislative. abbiamo proposto l'eliminazione di una norma un po' generica in quanto potrebbe rientrare tra le coperture già previste dalla disciplina contabile, ma soprattutto perché intervenire su quei parametri intervenire su quei parametri significa inasprirli, correndo il grave rischio di ricorso a risparmi incerti per coprire oneri certi. Quante volte la Commissione bilancio ha fatto i conti con la propria responsabilità proprio su questo terreno. L'altro emendamento è riferito all'aspetto informativo. È certamente positivo aver previsto nel DEF una specifica indicazione della spesa per interessi che lo Stato sostiene per aver sottoscritto strumenti finanziari derivati - è una battaglia antica, un'attenzione che era ma, a questo punto, perché non prevedere una simile indicazione per ogni sotto settore della pubblica amministrazione e i possibili scenari che possono delinearsi? Così potremmo conoscere anche l'impatto di tutte le operazioni in derivati sottoscritte da soggetti pubblici. Come messo in rilievo da una importante indagine conoscitiva del Senato della scorsa legislatura, l'impatto sulla finanza pubblica dei derivati sottoscritti dagli enti locali è tutt'altro che irrilevante. Il nuovo assetto contabile, quindi, sembra delineare regole adeguate a una necessaria revisione della precedente disciplina contabile in linea con le sempre maggiori pressanti esigenze, anche europee, di contenimento della spesa e del debito pubblico. Concludo, signora Presidente, dicendo che personalmente ritengo che il nuovo assetto contabile presenti nel suo complesso alcuni aspetti che meritano certamente un successivo approfondimento. Penso - ad esempio - al rapporto centro-periferia, forse ancora sbilanciato e con grandi margini di miglioramento, oppure - tanto per rimanere alla tematica della copertura delle leggi di spesa - alla soppressione dell'attuale articolo 11, che prevedeva anche la copertura degli oneri correnti recati dall'attuale legge di stabilità. la necessità di evitare la cosiddetta dequalificazione della spesa comporta che da qualche parte venga espressamente enunciato il divieto di peggiorare il saldo di parte corrente nel corso dell'esame parlamentare. Se il nuovo assetto contabile deve rappresentare un passo ulteriore in termini di garanzia di trasparenza e conoscibilità delle scelte compiute dall'azione pubblica, penso che le due questioni cui ho accennato possano e debbano trovare spazio nel dibattito e nei lavori parlamentari. La prima è complessa e ha bisogno di verifiche e approfondimenti; la seconda, invece, è necessario che la si affronti al più presto, sin dal prossimo ottobre. Speriamo e contiamo che l'introduzione del cosiddetto bilancio di genere, che

Signora Presidente, il disegno di legge, che oggi esaminiamo con parecchia fretta, reca alcune modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge rinforzata n. 243 del 2012. L'obiettivo di questa legge di iniziativa parlamentare è di modificare la meglio conosciuta legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, con il disegno di legge in esame si intendono unificare la legge di stabilità e la legge di bilancio in un unico provvedimento, unitamente ai relativi contenuti, nonché intervenire sul ciclo e sugli strumenti di programmazione finanziaria e sui tempi di presentazione dei documenti a essi annessi. In via definitiva, lo scopo principale che si intende perseguire è introdurre come obiettivi di programmazione economica - gli obblighi derivanti dalla citata legge rinforzata, apportando un ulteriore rafforzamento dei vincoli derivanti dal *fiscal compact*, per il quale il Movimento 5 Stelle ha sempre mostrato la sua forte disapprovazione. Per noi è fondamentale affermare la nostra contrarietà al legame stretto che viene istituito tra la legge che definisce i criteri e le modalità con cui costruire il disegno il disegno di legge di bilancio e la legge che ne detta invece gli obiettivi principali e i vincoli, ai quali siamo sottoposti per via dell'adesione a trattati sovranazionali, drammatiche i cittadini ignoravano. Questo è un aspetto che avremmo voluto fortemente evitare, anche alla luce del fatto che i nuovi strumenti di contabilità vengono condizionati ai famosi vincoli europei che vacillano ogni giorno di più e che osserviamo ciecamente senza alcuna considerazione del benessere collettivo, dei costi ambientali e soprattutto sociali. quali il BES (benessere equo e sostenibile), che contiene al suo interno indicatori che tengono conto dei fattori sociali, ambientali e di qualità della vita e della salute dei cittadini, potrebbe servire - appunto - per cambiare rotta. Si fa sempre più pressante la necessità di intraprendere una nuova direzione, la più ottimale possibile, che non solo tenga conto della necessità di perseguire la formula magica del PIL, ma che si avvicini di più ai reali bisogni di tutti noi. Per questo motivo, non mi stancherò mai di dire che, nella programmazione dei passi che un buon Governo intende realizzare, si dovrebbe iniziare a considerare gli indici del benessere equo e sostenibile, che andrebbero utilizzati quali parametri di riferimento, alla pari del PIL.

Anche questo modo di operare - un esame veloce e frettoloso - dimostra come questa maggioranza non sia disponibile a confrontarsi e a trovare convergenze significative, nonostante si tratti soprattutto di questioni relative alle regole. Per far funzionare un Parlamento, bisogna essere in due: una maggioranza e un'opposizione. Occorre che la maggioranza sia una libera intesa di donne e uomini non solo tolleranti, ma inclini alla discussione. La maggioranza, invece, si crede infallibile solo perché ha, dalla sua, l'argomento schiacciante del numero e pensa che basti l'aritmetica a conferirle il diritto di seppellire le opposizioni.

La barriera tra cittadino e istituzioni può e deve essere superata e se esiste ancora, la colpa va addebitata all'incapacità delle istituzioni, all'incuria dei governanti e a una precisa volontà politica. pensiero con le seguenti parole, non mie, ma a me molto care: «Il sogno è che la democrazia diretta si affermi e che il Movimento 5 Stelle, raggiunti i suoi obiettivi, non abbia più ragione di essere.

Grazie, Presidente. il provvedimento in esame è stato approvato alla Camera dei deputati a grande maggioranza, segno che, quando si vuole, le regole possono essere discusse e condivise anche con le opposizioni.

La drammatica fase economica in cui si trova il Paese impone regole più strette, efficaci e cogenti per tenere sotto controllo la situazione. Il pareggio di bilancio è ancora un miraggio, nonostante i proclami del Governo, e il debito pubblico galoppa verso traguardi impensabili e insostenibili. Il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio e i contenuti del DEF, che devono essere informazioni di dettaglio, le più puntuali di spesa, è quindi una necessità, altrimenti tutto quello che facciamo diventa carta straccia. I risultati delle politiche di entrata e le previsioni di spesa sui settori più importanti della vita del nostro Paese pubblico impiego, protezione sociale, sanità, debito delle pubbliche amministrazioni e spesa per interessi - debbono essere chiari, inconfutabili e indiscutibili. Sottolineo due buone cose contenute nel provvedimento, con riferimento alla legge di spesa, che mi stanno particolarmente a cuore. Finalmente viene esclusa la possibilità il Governo di utilizzare la quota dell'otto per mille e del cinque per mille del gettito IRPEF, devoluto alla diretta gestione statale, per finalità diverse

Con l'otto per mille e con il cinque per mille sono state risolte varie problematiche, perché la legge prevedeva l'utilizzo di quelle somme per salvare beni culturali in situazioni di grave degrado, per le calamità naturali, per la fame nel mondo, per l'assistenza

Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi senatrici e senatori, con questo provvedimento si porta a compimento il processo di riforma dell'ordinamento contabile contabile avviato, dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo, con la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e poi proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012. del 2012. Sempre in questi giorni la Camera è chiamata ad approvare l'altro pilastro della riforma, ovvero quello sulle nuove regole per i bilanci di regioni ed enti locali, che ha già ricevuto l'approvazione del Senato. Come è stato ben illustrato nella relazione del senatore Azzollini, il provvedimento in approvazione si sostanzia di un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, e che vi apporta numerose modifiche e integrazioni, così come aggiunge ulteriori articoli. articoli. Innovazioni rilevanti vengono apportate in relazione alla programmazione delle risorse, al monitoraggio degli obiettivi di spesa da conseguire, ampliando, al contempo, i margini di flessibilità di bilancio. avviene sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che nella fase gestionale. Questi margini di flessibilità sono funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e una migliore programmazione delle risorse, oltre che

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla riforma - come è stato già ricordato dal relatore - vi è una manovra annuale che sarà definita con un unico provvedimento, composto da una prima parte di disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, ovvero gli attuali contenuti della legge di stabilità, e una seconda parte di natura tabellare che assorbe la vecchia legge di bilancio. di bilancio. Queste nuove regole consentiranno l'impostazione e la gestione di una manovra di bilancio più agile e moderna, in linea con quanto viene fatto in altri Paesi avanzati, - altro aspetto importante - sarà in grado di superare quella frammentazione di innumerevoli micronorme che - come sappiamo bene - hanno caratterizzato finora questo provvedimento. In tema di modifiche al processo di formazione del bilancio dello Stato, il perno della riforma è rappresentato dal nuovo dispositivo che collega in modo rigido la decisione di bilancio all'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché - come avviene oggi - alla loro variazione al margine. Ciò renderà strutturale e non più episodica la manovra di revisione e ricomposizione della spesa, la cosiddetta *spending* *review*. Come evidenziato da numerosi contenuti del disegno di legge, credo sia da sottolineare come in questo modo potrà essere rafforzato un approccio di politica economica cosiddetto *top down*, dall'alto verso il basso; un processo di formazione, cioè, che innova profondamente rispetto all'esistente e che gioverà sicuramente all'efficacia della strategia complessiva di politica economica da formulare. Questa maggior efficacia è altresì confermata dal fatto che si potranno superare le attuali criticità, in particolare introducendo specifici incentivi per riconsiderare la spesa storica, oltre che gli incrementi marginali. Come ho detto, si potrà così facilitare e rendere continuativo il percorso di ricomposizione e di revisione della spesa.

A tal fine, è da sottolineare come positiva la previsione della definizione su base triennale degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero; una programmazione in coerenza con gli obiettivi che vengono fissati per l'intera amministrazione pubblica sia nel DEF che nella manovra complessiva di bilancio. Allo stesso tempo, si prevede che, in vista dell'approvazione del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e i singoli Ministri di settore possano siglare dei veri e propri accordi su modalità e termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. altro dato da sottolineare è che, con questo provvedimento, cambierà la fisionomia anche del Documento di economia e finanza. in poi, contenere informazioni di dettaglio su risultati e previsioni triennali dei conti dei principali settori di spesa, in particolare con riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale, alla sanità, nonché informazioni e previsioni sul debito e sul relativo costo medio.

parlamentare; nonché il fatto che è stato reso trasparente il raccordo tra le previsioni di bilancio e l'insieme delle autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto.

soprattutto per la possibilità di superare l'approccio che vedeva la Ragioneria generale dello Stato iniziare quel provvedimento attraverso l'emanazione di una circolare con cui si invitavano i Ministeri a trasmettere le proprie valutazioni per la formazione complessiva del bilancio. Il superamento di tale procedura, credo, consentirà altresì di dare maggiore organicità, oltre che flessibilità, all'azione dei Ministeri di settore rispetto agli obiettivi a essi conferiti. Allo stesso modo, credo possa essere sottolineata una maggiore forza proprio nella considerazione del complesso delle richieste di dotazione finanziaria, rispetto alle varie funzioni da svolgere. È già stata sottolineata la novità del calendario, ovvero la possibilità che entro il 27 settembre venga presentata la nota di aggiornamento al DEF e poi il Parlamento e la Commissione europea, oltre che l'Eurogruppo, riceveranno entro il 15 ottobre il documento unificato di bilancio. Anche io sottolineo con favore l'introduzione di nuovi indicatori per la valutazione di impatto delle norme,

per ogni Paese sia per la sua comparabilità nel tempo, sia per la sua comparabilità a livello internazionale. In questo caso si tratta di integrare e in qualche modo completare le indicazioni di carattere macroeconomico, con una programmazione che possa tener conto anche di altri aspetti importanti. Naturalmente, bisognerà valutare con attenzione il fatto che questi indicatori hanno tempi di misurazione diversi e, soprattutto, rapporti di causa-effetto diversi. Questo naturalmente non ci impedisce di sottolineare con favore il fatto di avviare una sperimentazione di questo genere.

In primo luogo, con l'unificazione in un solo strumento legislativo della legge di stabilità e della legge di bilancio, si creano le condizioni per il superamento del vizio fondamentale

trascurandone completamente la parte prevalente. In secondo luogo, questa decisione consente di valorizzare pienamente gli effetti sul bilancio del mutamento non della legislazione, ma dei comportamenti e delle attività amministrative, fino ad oggi completamente trascurati nella decisione di bilancio stessa, a tutto vantaggio dell'innovazione legislativa, ovvero del contenuto dell'attuale legge di stabilità. Attraverso l'unificazione di legge di stabilità e legge di bilancio, noi ci mettiamo - questo è il punto ed è un salto di qualità enorme della decisione di bilancio - sulla strada che sulla strada che può finalmente portare al cosiddetto bilancio a base zero, che può mettere su gambe solide la revisione della spesa, fino ad oggi ostacolata da una decisione di bilancio che agisce nella logica meramente incrementale, cioè delle variazioni ai margini della componente storica del bilancio stesso. In questo modo, il bilancio pubblico italiano - l'unico, nel contesto europeo, a mantenere ancora questa caratteristica - perde il carattere di legge fotocopia della legislazione vigente di entrata e di spesa, per assumere quello di una legge che contiene scelte di politica economica e fiscale funzionali al conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza, a loro volta coerenti con quelli definiti in sede europea nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle politiche economiche e fiscali che spettano agli organismi europei. Ecco, sul rapporto tra decisione e gestione di bilancio a livello nazionale e coordinamento delle politiche fiscali ed economiche nella dimensione europea, è emerso l'unico elemento di profonda distinzione politica tra

sia in Commissione sia qui in Aula, emendamenti volti a cancellare dalla legge al nostro esame qualsiasi riferimento all'ordinamento europeo; in Aula, ad esempio, c'è l'emendamento 1.18 che ha questo carattere. È una scelta assolutamente legittima, e di enorme rilievo per il presente e per il futuro del Paese, di cui vorrei sottolineare appunto l'importanza politica. [**Presidenza abbiamo chi vuole cambiare il segno della politica economica e fiscale prevalente in Europa (prevalente nel recente passato e in larga misura anche nel presente), ma ritiene indispensabile e assolutamente irrinunciabile iscrivere le scelte di politica economica e fiscale nazionale nel quadro, da rafforzare e da approfondire, di una vera e propria politica economica e fiscale fiscale europea, ritenendo che, fuori da questo contesto, ci siano solo impotenza e marginalità. Dall'altra c'è chi rifiuta la dimensione europea come tale, in una logica sovranista che sembra ritenere che ci sia salvezza per i singoli Stati europei, quindi anche per l'Italia, fuori dalla dimensione europea e infatti sostiene scelte, come ad esempio che potrebbero determinare la disgregazione della dimensione europea come dimensione capace di agire nel contesto dell'economia globale da protagonista. Ecco, questa distinzione profonda è l'unica davvero politicamente rilevante ad essere emersa da una discussione, prima alla Camera e adesso al Senato, che per il resto, sulle scelte che riguardano la tenuta della contabilità nazionale e la decisione di bilancio, ha fatto segnare una larga convergenza *(Applausi

è stata di privilegiare l'esigenza dell'immediata entrata in vigore delle norme che, come concordemente abbiamo visto, è particolarmente sentita, rispetto a un miglioramento del testo che pure, a mio avviso, è necessario e che sarà possibile, tant'è che il relatore ha presentato alcuni ordini del giorno

dopo un'attenta considerazione si è ritenuto di poter in questo momento soprassedere, attraverso ordini

1.2, anche perché la Presidenza del Consiglio dei ministri è sicuramente già compresa nella nozione di «pubbliche amministrazioni». Naturalmente, al parere contrario è associato prima, ove i senatori presentatori volessero, un invito al ritiro, anche in ragione del tipo di parere che sto

l'accesso del Parlamento alle banche dati in generale deve essere regolamentato, come un testo normativo, dai Regolamenti parlamentari. Anche in Commissione abbiamo ritenuto ultronei questi emendamenti, ma nel contempo faccio appello alla Presidenza perché con i Regolamenti parlamentari si

è utile che il Parlamento nel suo complesso ne possa usufruire secondo i Regolamenti, così come previsto dalla normativa precedente. Per questo motivo esprimo parere contrario

1.12 perché la diffusione dei dati non mi pare assolutamente conferente con l'attuale sistema normativo di presentazione del bilancio.

dell'apprezzamento che la senatrice Bonfrisco ha rivolto al testo di legge anche perché ella è stata particolarmente interessata a questo problema, ma non è in questa norma ordinamentale o nel bilancio dello Stato che possono essere essere espressi dati così tecnici che invece vanno trattati nelle sedi opportune. Riconosco, naturalmente,

prima alle Camere piuttosto che agli organi di stampa, per una ragione ovvia di

Ciò significa che abbiamo fatto in termini di trasparenza un salto molto importante di qualità proprio in queste ore.

del grande pericolo all'interno dei bilanci degli Stati (non solo il nostro) e di altre istituzioni finanziarie quanto mai importanti come quelle bancarie e quindi degli effetti non non noti e così poco conosciuti, anche in virtù della loro natura, dei derivati che potrebbero continuare a nascondere perdite nell'ammontare degli interessi sul debito che ancora non conosciamo.

abbiano inteso sostenere l'azione del Governo affinché questo dato sia reso noto il più possibile. Ricordo però, solo per cronaca, come, qualche tempo fa, una richiesta del Parlamento di conoscere gli effetti prodotti dai derivati sul bilancio dello Stato sia stata respinta dal Governo, che ha inteso impedire l'accesso agli atti ai parlamentari. Vorrei quindi tornare a richiamare l'attenzione del Governo affinché in questa fase la trasformazione dell'emendamento 1.23 in un ordine del giorno possa costituire comunque l'inizio di un percorso assai più positivo e trasparente tra Governo e Parlamento sulla questione dei derivati. Non penso ci siano Governi che possano o vogliano nascondere questo dato; penso che un ordine del giorno indichi una volontà precisa del Parlamento e che questo Governo abbia, secondo me, tutto l'interesse ad accoglierlo.

sono d'accordo con il relatore. Faccio notare, peraltro, che il testo, accogliendo un emendamento presentato alla Camera, quindi un'iniziativa parlamentare, già contiene la scelta di evidenziare (laddove si affronta il tema dell'evidenziazione della spesa per interessi) separatamente e distintamente la spesa per interessi da

la seconda parte, invece, non sarebbe accolta dal Governo se la proponente insistesse sulla sua presenza nel testo dell'ordine del giorno.

la valutazione cosiddetta degli scenari probabilistici è quella che indica l'Unione europea per poter analizzare con precisione il peso, anche nascosto, degli strumenti di finanza derivata rispetto a quel costo atteso (il *mark to market*, come lo definisce il linguaggio finanziario) il quale, oltre che della probabilità di perdite e dei rischi connessi a tali strumenti, si occupa anche della proiezione futura. Chiedo che l'ordine del

con questo emendamento, al di là della sua formulazione tecnica che riprende esperimenti che già erano in vigore (e infatti nell'ordine

della Camera è stato ben fatto: ha già introdotto alcuni vincoli rispetto all'attuale formulazione della clausola di salvaguardia. Ma il problema che ho posto è che, trattandosi in questo caso di norma ordinamentale, dobbiamo avere l'ottica del lungo periodo, nel quale il problema del debito

in altri provvedimenti si introducano norme più stringenti nel caso di disallineamento, nello stesso esercizio, in particolare, tra onere e copertura. La proposta formulata attiene a fondi negativi, che sono una tecnica

alla reintroduzione dei fondi negativi. Non abbiamo il tempo per approfondire l'argomento, ma la sostanza è che storicamente abbiamo avuto due forme di clausole di salvaguardia

si dice in partenza che 50 di quei 100 non potranno essere effettivamente spesi, a meno che non si verifichino determinate condizioni. Il fondo negativo voleva dire un freno alla spesa che, naturalmente, in corso d'anno introduce un'enorme incertezza sulle dimensioni e sulla qualità della spesa stessa. Abbiamo poi sostituito i fondi negativi con le attuali clausole di salvaguardia che - detto in un linguaggio da bar

regole e delle condizioni di bilancio. La soluzione che abbiamo adottato nella legge a me sembra, con larghissimo consenso, superare entrambe queste tipologie per introdurre un vincolo politico fortissimo sul Governo

Signor Presidente, comprendo la *ratio* con cui il senatore Azzollini, nella sua veste di relatore, esprime un parere contrario. So che non è nel merito, ma attiene alla parte formale...

compatibile con la legge generale dell'ordinamento di contabilità. Per questo motivo, sono contrario

oggi necessario agli enti locali per la progettazione di quelle infrastrutture che vediamo non partire mai nonostante i grandi sforzi che i Governi compiono, è al centro di questa sollecitazione che pongo al rappresentante

il Fondo rotativo per la progettazione è istituito con la legge n. 549 del 1995, presso la Cassa depositi e prestiti. È cioè un fondo che già esiste e che è stato molto poco utilizzato.

con la valorizzazione immobiliare si sono realizzate tante cose in questo Paese. Quindi, forse è giusto che i Comuni, le Regioni e anche i Ministeri possano avere a disposizione un fondo di rotazione che poi viene rimpinguato all'atto della concessione del finanziamento. Utilizzarlo anche per le valorizzazioni

della comprensibilità di tutti gli aggregati a supporto della manovra complessiva. l'introduzione degli indicatori di benessere e il superamento di una certa rigidità, che fino ad ora ha fatto percepire le manovre complessive come

Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando riveste un'importanza enorme. Esso rappresenta un ulteriore tassello di quel processo di modificazioni alla legge di contabilità iniziato nel 2009 con la legge n. 196 e poi continuato con la legge n. 243 del 2012. Si tratta di un provvedimento che rappresenta anche lo strumento di cui ci serviamo per attuare l'articolo 81 della Costituzione, quello sul pareggio di bilancio, che tante polemiche ha periodicamente suscitato. Una norma, come si è detto tante volte, inserita in Costituzione per imposizione dell'Unione europea o per supina acquiescenza da parte nostra nei confronti dei *Diktat* provenienti da Oltralpe. Ma comunque sia, vincoli o no, il valore essenziale che un Paese serio deve perseguire è quello di avere i conti in ordine e a posto e, per far questo, non bisogna certamente attendere che qualcuno venga a dircelo: deve essere un'esigenza nostra, una responsabilità nostra. Cosa diversa è invece sentire l'esigenza che il bilancio goda di una certa equilibrata e sana capacità di essere flessibile, soprattutto per fronteggiare imprevedibili fasi economiche di crisi, dove l'eccessiva rigidità delle regole di bilancio finisce per diventare dannosa e paralizzante per qualunque amministrazione. Ebbene, questo provvedimento ci consente di fare l'una e l'altra cosa, perché l'articolo 81 non prevede un pareggio in senso stretto, ma l'equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto delle congiunture avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. E dobbiamo intenderci sul fatto, cari colleghi, che in un Paese come il nostro, caratterizzato da un elevato debito pubblico, è cosa necessaria avere un bilancio in equilibrio e dei conti seri, a meno di voler convivere con il rischio angosciante della della possibilità di *default*. Del resto, abbiamo visto come in questi tre anni la flessibilità non è stata impedita, anzi è stato spostato, con tre provvedimenti distinti, il pareggio strutturale di bilancio di tre anni, dal 2016 al 2019, seguendo le norme dell'articolo 81 e senza che l'Unione europea osservasse alcunché. Altra cosa è poi interloquire in maniera diversa e più efficace con l'Unione europea, affinché le politiche europee segnino un concreto cambio di passo, specie in questo momento in cui le istituzioni europee vivono un momento di forte crisi e di mancanza di credibilità per larghe fasce di cittadini. Occorre quindi rivedere i programmi di *austerity*, puntare di più sull'occupazione e sullo sviluppo e superare la mera unificazione monetaria, per approdare a una integrazione politica più forte, più condivisibile e più vivibile. Ma torniamo al merito. Questo provvedimento è teso essenzialmente a semplificare la legge di bilancio, facendo venire meno la legge di stabilità, con tutte quelle previsioni fuori sacco che annualmente si traducevano in un vero e proprio assalto alla diligenza, con le norme più disparate e varie racchiuse in un unico, caotico calderone di disposizioni, il cui filo conduttore era praticamente impossibile da individuare. Adesso il contenuto dell'attuale legge di stabilità sarà assorbito dalla legge di bilancio, che sarà redatta solamente con le misure volte a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, ovverosia il DEF la relativa Nota di aggiornamento. Ci sembra un buon esempio di semplificazione e di trasparenza, nella ricerca del miglioramento della regolazione contabile, che non deve servire soltanto a chi ne fruisce nel momento contingente, ma aspira a porsi come modello durevole di riferimento anche per chi verrà a governare e a legiferare dopo di noi. Infatti questo provvedimento reca in sé degli effetti importanti di tipo politico, che si traducono principalmente nell'intelligibilità dei dati, che quindi potranno essere compresi non solo dal legislatore, ma da tutti coloro che vorranno appassionarsi alla contabilità pubblica. Questo comporterà quindi fornire con grande trasparenza ai cittadini elementi di valutazione per poter giudicare le scelte di politica economica fiscale, ma anche altre dinamiche legate alle decisioni politiche. Questo è un elemento importantissimo che non deve essere sottovalutato e anzi ne va enfatizzata la presenza,

viene concentrato in una sola legge e viene superata la separazione tra legge di bilancio e legge di stabilità e quest'ultima viene assorbita nella legge di bilancio. In secondo luogo, viene potenziato il bilancio di cassa, dal momento che lo si allinea meglio con la competenza, rendendolo più razionale inoltre, viene superata la possibilità degli interventi microsettoriali e localistici. Ancora, il testo fornisce un maggiore accesso ai dati, anche ai *software* utilizzati per la gestione dei dati da parte del Governo ai fini della delineazione della manovra di finanza pubblica. Tutto questo è positivo perché renderà più comprensibile anche ai cittadini il meccanismo di approvazione del bilancio dello Stato. Vengono superate le rigide norme di salvaguardia, che in questi anni hanno generato problemi e polemiche, non nel senso che queste scompariranno del tutto, ma nel senso che saranno meglio definite e declinate. Questo è un aspetto positivo, perché vengano evitate spregiudicate manovre e manovrine dell'ultima ora, o automatici e insopportabili aumenti della pressione fiscale. È previsto un coinvolgimento maggiore del Parlamento, anche se questo particolare aspetto dovrebbe essere ancora migliorato. In ogni caso, il Documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri viene inviato contestualmente sia a Bruxelles che al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno e questo depone per l'affermazione di un sussulto di dignità nei confronti della Commissione europea, cosa che in questi anni, a mio giudizio, è mancata. Una cosa importante e più che corretta, perché va nella direzione del rispetto delle scelte dei cittadini è il fatto che viene esclusa la possibilità di utilizzare i fondi dell'8 per mille e del 5 per mille per esigenze straordinarie di finanza pubblica. Ancora, nel testo troviamo una novità che ci sentiamo di apprezzare molto e cioè l'inserimento dell'utilizzo degli indicatori di benessere ecosostenibile (BES), nella valutazione e nell'orientamento delle scelte e delle politiche di bilancio. Si tratta di una cosa assai importante che vogliamo sottolineare, perché è un elemento significativo di innovazione, che ci dice che non basta il PIL per comprendere quale sarà il reale impatto che le manovre economiche determineranno nel tempo e nella nostra società, ma occorre far riferimento, appunto, ad altri indicatori come la qualità sociale o la sostenibilità ambientale. Certo, siamo ancora un po' lontani dall'obiettivo della realizzazione del cosiddetto bilancio ambientale, ovvero l'utilizzo di una modalità e di una logica nuova che permetta di valutare le ricadute, dal punto di vista della sostenibilità e della qualità della vita, della totalità degli interventi posti in essere dall'amministrazione pubblica, dal momento che la sostenibilità va considerata quale elemento trasversale a tutte le scelte politiche che possano essere operate. Ma in ogni caso, al momento ci accontentiamo. Alla fine, al di là dei tecnicismi, a questo servono il bilancio e la contabilità pubblica: incidere positivamente nell'esistenza delle persone, garantirne il diritto al lavoro, tutelarne i diritti civili e la salute, operare per il benessere di ognuno e rendere questo nostro Paese ancora capace di futuro. Se tutto questo non è percepibile e non impatta in maniera concreta sulla vita delle persone, sarà vano ogni nostro tentativo di allenarci su improbabili funambolismi tecnici e legislativi. Forse potremo creare qualche effetto speciale, buono a stupire noi stessi, ma non avremo cambiato di una virgola la quotidianità delle persone, che oggi è troppo spesso faticosa e incerta e ci chiama a nuove responsabilità. Con questo spirito di apprezzamento del lavoro fatto, e di auspicio per ulteriori, futuri miglioramenti, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie.

di bilancio si fa un passo in avanti, anche sensibile, e si introducono alcuni concetti che prima erano assolutamente assenti nella manovra: quello sul benessere ecosostenibile abbia un valore particolare. Concludo con la speranza che questa forma che noi stiamo adottando serva anche a qualificare meglio l'azione del Parlamento sul piano della programmazione economica. mentre sulle scritture di bilancio, sul contenimento della spesa e sulla trasparenza - lo voglio dire - delle scritture contabili qualche passo in avanti è stato fatto, sui temi della programmazione economica anche il Parlamento e le Commissioni preposte a questa funzione, insieme ovviamente alla responsabilità prima del Governo, non sono ancora all'altezza del bisogno.

in quell'azione riformatrice a livello politico e legislativo che questo Governo, con il contributo imprescindibile della forza che rappresento, sta portando avanti in materia di regole di bilancio e contabilità. Gli interventi di questo disegno di legge si innestano in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio, avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, modificativa dell'articolo 81 della Costituzione. In quell'occasione è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio, demandando a una successiva legge rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione e la definizione del contenuto della legge di bilancio. Tratteggiando un breve quadro di sintesi, ci troviamo di fronte a una fase di complessiva riforma del bilancio dello Stato, che risulta completata da altri tre provvedimenti: in particolare, la delega sul completamento della struttura del bilancio *ex* articolo 40 della legge di contabilità, su cui abbiamo espresso il parere nel febbraio 2015, i cui contenuti sono stati trasfusi nel decreto legislativo n. 90; la delega sul potenziamento della funzione di bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42 della legge di contabilità; il disegno di legge in corso di esame alla Camera, con il quale si modificano gli equilibri dei bilanci per Regioni ed enti locali, per rafforzarne il ruolo di cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento e incoraggiare una gestione più efficiente Il disegno di legge in esame, che procede parallelamente con quello appena citato, assume una valenza semplificatoria e di razionalizzazione delle procedure per la formazione del bilancio dello Stato: si prevede, infatti, l'integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale (disegno di legge di bilancio e di stabilità) e si dispone il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. Inoltre, si interviene sul documento programmatico di bilancio, disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento che non prevede, al momento, tale trasmissione al Parlamento. Sui contenuti del DEF si interviene poi mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del documento quelli riferiti al BES, ossia al benessere equo e sostenibile. Una modifica rilevante prevista all'articolo 1 del provvedimento attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità: si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni: la prima, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è, invece, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Altro elemento centrale della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Si dispone l'eliminazione di tali clausole con l'introduzione di una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi.

concertati con il Governo, in parallelo nelle due Commissioni; li abbiamo discussi ovviamente prima alla Camera e poi al Senato, ma in forma sostanzialmente congiunta, in modo da arrivare oggi a un testo Da senatore del Partito Democratico vorrei invece esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo su un provvedimento di straordinaria importanza, che è stato già definito dal collega Guerrieri Paleotti come una riforma strutturale ed è tale perché completa un trittico

una riforma strutturale della quale è difficile sopravvalutare l'importanza per il Paese se solo si tiene conto del fatto che, grosso

della ricchezza che producono gli italiani viene in qualche modo gestita della spesa pubblica, dallo Stato, ed è assolutamente chiaro che le modalità di gestione e di governo di questa spesa sono essenziali

Una ricchezza del Paese, che ammonta a 800 miliardi su 1.600 miliardi di prodotto interno lordo gestiti dallo Stato, che non riesce a produrre

Naturalmente questo risultato, che certamente credo non sia soddisfacente per nessuno in quest'Aula, ha a che fare con la politica, con gli indirizzi politici di questo e quel Governo e di ciò discutiamo in altra sede tutti i giorni,

Camera e Senato, nell'Aula di Montecitorio e oggi nell'Aula di Palazzo Madama - una larga maggioranza ha detto che, ferme restando le differenze che abbiamo dal punto di vista politico e problematico, vogliamo modernizzare insieme lo strumento di governo del bilancio e quindi di quella metà della ricchezza degli italiani che in qualche modo fa riferimento allo Stato. Non torno sui contenuti di questa riforma; è già stato fatto ampiamente dal relatore Azzollini, che ringrazio, come sempre, per la puntualità, la disponibilità e l'intelligenza politica con cui ha accompagnato questo percorso; l'hanno detto il vice ministro Morando

che ci consente di evitare questo rito dell'assalto alla diligenza che ogni anno si ripete in Parlamento, peraltro su una quantità minima di risorse rispetto all'universo del bilancio. C'è finalmente la possibilità di intervenire sul bilancio nel suo insieme, anche attraverso l'azione amministrativa, non solo quella legislativa, in modo da rendere effettiva la revisione della spesa e quindi l'uso ottimale delle risorse pubbliche.

l'introduzione di un elemento qualitativo della valutazione dell'uso della ricchezza pubblica, rappresentato, appunto, dagli indicatori di benessere equo e sostenibile. Vorrei rapidamente toccare due punti politici che mi sembrano di assoluto rilievo. Il primo riguarda il nesso tra questa riforma e la riforma dell'articolo 81 della Costituzione che abbiamo approvato nella scorsa legislatura, nel 2012. Spesso si sente dire che con il nuovo articolo 81 Governo e Parlamento si sono legati le mani, che abbiamo vincoli maggiori rispetto alla possibilità di usare il bilancio in chiave espansiva. Ciò che stiamo votando oggi è la prova del contrario: stiamo votando una legge di contabilità che consente quella flessibilità, attenta al ciclo economico, che il vecchio articolo 81 della Costituzione non consentiva e che, invece, il nuovo articolo 81 prevede e disciplina in maniera seria e rigorosa. quindi, uno strumento di contabilità pubblica legato alla nuova Costituzione, dipendente dal nuovo articolo 81 introdotto nella Costituzione, che consente alla politica - alla buona politica - di fare davvero il suo mestiere, quindi di usare le risorse in modo oculato nelle fasi espansive, per produrre quel*surplus* che, poi, nelle fasi recessive del ciclo può essere utilizzato per sostenere la domanda. L'ultimo punto, quello sul quale si è marcata una distinzione e una differenza, in particolare con i colleghi del Movimento 5 Stelle, riguarda il rapporto con l'Europa.

il nostro governo delle risorse pubbliche con le decisioni che vengono assunte insieme a livello europeo. Non è una devoluzione di sovranità, ma una condivisione della sovranità che abbiamo deciso di mettere insieme con gli altri che con noi condividono l'avventura straordinaria della moneta unica e della costruzione dell'Europa politica. Oggi noi siamo insoddisfatti di come funziona Oggi noi siamo insoddisfatti di come funziona l'Europa, ma - attenzione - non perché si debba e si possa tornare indietro a più sovranità dei singoli Stati e delle singole Nazioni, ma perché si deve costruire insieme un patto un patto che sia non solo di stabilità, ma anche di crescita. Questo è l'elemento di difficoltà del nostro sistema. Qualche anno fa si diceva accanto al *fiscal compact* ci doveva essere un *growth compact*, cioè un patto per la crescita. Il problema non è rimettere in discussione il Patto di stabilità, e quindi anche il *fiscal compact*, ma è come accompagnare al *fiscal compact*, cioè ad un patto della serietà fiscale (che deve ridurre l'indebitamento, ovvero lo spreco delle risorse pubbliche), un patto che sia davvero per la crescita

e divide lo schieramento politico italiano, e non solo italiano. In questo senso, l'approvazione della riforma della legge di contabilità ci consente di fare un deciso passo in avanti.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, anticipo subito che il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente all'approvazione di questo provvedimento. Oggi stiamo esaminando le regole del gioco, i precetti per scrivere nel modo più appropriato i numeri della contabilità pubblica. Queste sono decisioni che si prendono tutti insieme, tanto che alla Camera il nostro Gruppo ha già partecipato all'approvazione di questo provvedimento. Del resto, qui a Palazzo Madama abbiamo fatto parte dello schieramento trasversale che ha firmato il disegno di legge del presidente la legge di contabilità del 2009 viene nuovamente ritoccata in attuazione della legge rinforzata n. 243 del 2012, conseguente alla novella costituzionale dell'articolo 81. L'obiettivo è innanzitutto quello di adeguare il procedimento contabile al nuovo contesto costituzionale. L'introduzione di una legge unica, che ne sostituisce due, integrando nella legge di bilancio tutte le previsioni della legge di stabilità, dovrebbe servire a semplificare il quadro della finanza pubblica. Sto usando il condizionale, perché quest'anno il Governo varerà la prima nuova legge di bilancio e solo dopo potremo trarne, tutti insieme, le conseguenze. Valuteremo, quindi, il suo funzionamento, la tecnicità; valuteremo se le norme ora al nostro esame necessiteranno di un un eventuale tagliando. Siamo comunque sulla strada che porta a un provvedimento che va a esporre e rendere più comprensibile, all'interno delle due sezioni della legge di bilancio, le scelte di politica economica prese ogni anno dal Governo, entro il 20 di ottobre. oltre a innovare nel metodo, vi sono anche alcune novità nelle date, nel calendario della redazione e presentazione dei documenti di economia e finanza da parte del Governo alle Camere e in Europa. Si sta andando incontro a un nuovo scadenziario e a un nuovo elenco degli strumenti di politica economica, che dovrebbero essere più adatti al nuovo quadro di regole costituzionali. Vero è che si cerca di incrociare le esigenze del bilancio con le metodologie attraverso le quali l'ISTAT comunica le scelte italiane di politica economica all'Europa. Anche per il Documento di economia e finanza si prevede un'integrazione con informazioni di maggiore dettaglio sulla spesa, ma si attende anche una migliore definizione dei debiti delle pubbliche amministrazioni e del loro onere. Sarà utile conoscere anche il valore della spesa per interessi messa in relazione agli strumenti finanziari derivati, considerate le situazioni che si sono purtroppo registrate in tal senso negli ultimi anni per errori politici, ma anche tecnici. Su questo tema un maggiore controllo del Parlamento non può che essere utile, oltre che ragionevole. Entra in campo anche il nuovo indicatore del benessere equo e solidale (BES), definito il quale si dovrebbe procedere a politiche meglio finalizzate in campo sociale, che aumentino il *welfare* e riducano gli sprechi. Inoltre, con il disegno di legge al nostro esame viene eliminato il meccanismo delle clausole di salvaguardia sulle imposte e sulle accise (qualcuno stamattina diceva finalmente!). Esso viene sostituito da clausole sulla spesa, senza però garanzie sufficienti che queste non finiscano per ridurre il livello qualitativo dei servizi ai cittadini ovvero ne facciano crescere l'onere a diretto carico degli interessati. Noi restiamo da sempre a favore dell'individuazione di coperture certe, attraverso, per esempio, tagli ai tanti sperperi presenti in quell'area non trasparente che si colloca tra gli appalti, le gare pubbliche e la politica. Proprio per quanto detto, pur apprezzando la nuova forma della legge di contabilità, a noi rimangono ancora diversi dubbi. Sin dalla riscrittura della Carta costituzionale e della legge rinforzata nel 2012, infatti, si sarebbe dovuto assegnare un differente peso sopratutto alla tutela del contribuente; tutela che manca nella Costituzione, nella legge rinforzata e, di riflesso, anche in questo disegno di legge. Quando si tenne il dibattito sulle modifiche dell'articolo 81, tra le idee messe in campo, fu presentata anche quella di porre un tetto alla spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo. Allora non mancarono nemmeno proposte che intendevano fissare il limite massimo della pressione fiscale. Fu presente anche l'ipotesi di poter utilizzare l'indebitamento solo facendo ricorso a una maggioranza molto amplia - i due terzi di ogni Camera - che, quindi, vedesse anche le minoranze parlamentari concordi nel ricorso al *deficit*. Erano tutti indicatori che assegnavano al Parlamento il controllo della spesa pubblica. Si scelse, invece, la strada impervia dell'equilibrio di bilancio, che segnò un passo indietro rispetto alla previsione di scrivere nella Costituzione le parole: «pareggio di bilancio». Ora, su questi presupposti, noi riscriviamo la legge di contabilità senza assegnare alcuna tutela a chi tiene in piedi il Paese pagando le tasse. Sto pensando ai tanti lavoratori dipendenti che non possono sfuggire ai versamenti grazie alla figura del sostituto d'imposta, ma anche agli autonomi che si fanno carico di regole fiscali penalizzanti nei loro confronti, quali le minori detrazioni da lavoro, le imposte versate in anticipo sui redditi presunti e i maggiori adempimenti burocratici. Penso persino alle imprese che credono nel nostro Paese, le quali, con processi aziendali all'avanguardia, producono utili e pagano le tasse in Italia e non, magari, in Olanda. Dobbiamo rilevare, obiettivamente, che nei quattro anni di applicazione pratica del nuovo articolo 81 della Costituzione le finanze pubbliche non sono migliorate. Al contrario, il loro deteriorarsi è dovuto proprio al ricorso smisurato all'indebitamento. L'utilizzo di manovre in *deficit* ha avuto un impatto peggiore di quello che ebbe la famigerata sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, in conseguenza della quale presero il via le norme prive di copertura, che hanno dato la stura alla crescita del debito italiano. Il relatore, per curiosità, si chiamava Cassandro e, ironia della sorte, non seppe prevedere quali danni quella decisione della Consulta avrebbe creato alle finanze pubbliche negli anni a venire. Fino alla metà degli anni Sessanta il miracolo italiano si era basato anche sul rigore finanziario dei conti pubblici, che in quei tempi, quasi ogni anno, ci regalava persino un avanzo primario. Poi, dopo molti anni di crescita del debito e di mancata crescita dell'economia, nel 2012, anziché invertire il *trend*, si è fatto ricorso sistematicamente all'indebitamento, prima in presenza di cicli economici avversi e, poi, continuando anche quando ha soffiato il vento in poppa, donando una fase ciclica positiva all'economia. Questo ha portato allo *stock,* che ormai ogni anno cresce con un *record* storico in negativo (l'ultimo pari a 2.242 miliardi di euro). E vorrei ricordare, solo per lasciarlo alla memoria dei Resoconti, che il montante complessivo del debito era di 1.906 miliardi alla fine del 2011, quando cadde l'ultimo Governo eletto, quello di Silvio Berlusconi. La preoccupazione è che gli effetti sui conti pubblici si faranno sentire quando finiranno le cartucce del *bazooka* di Draghi e saranno probabilmente inservibili le ulteriori armi di politica monetaria a disposizione della Banca in questo momento storico italiano la crescita economica è zavorrata da una pressione fiscale che ha raggiunto livelli inaccettabili, proprio perché le manovre fatte a debito hanno sbagliato, secondo noi, la destinazione delle risorse, non hanno agevolato gli investimenti e hanno prodotto un erroneo ricorso alla leva fiscale. Quindi, non bastano gli annunci di riduzione di un punto della prima aliquota IRPEF, fatta trapelare da ambienti governativi; è necessario un autentico e ragionato *shock* fiscale, che al contempo consenta di allargare la base imponibile, fondandola su un PIL che cresca a ritmi elevati. In altre parole, occorre una riduzione fiscale importante e coraggiosa che inneschi accompagni la crescita, anziché frenarla. Se la nuova legge di contabilità che porta con sé la nuova legge di bilancio servirà a questo, sarà la benvenuta. In caso contrario, continueremo ad avere misure estemporanee, altri *bonus* da 80 o da 500 euro, *bonus* *bebè* o *bonus part-time*, altre manovrine senza cuore né coraggio, che gli italiani non meritano e che non produrranno nulla di buono per il nostro Paese.

finestra"). L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione. Con ricorso depositato il 29 gennaio 2016, il tribunale di Bergamo - sezione dibattimentale penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 settembre 2015, ha dichiarato che i fatti, oggetto di un procedimento penale, per i quali il senatore Calderoli è stato chiamato a rispondere, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993; nella stessa seduta l'Assemblea ha invece ritenuto non applicabile la prerogativa in questione alla fattispecie di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 maggio 2016, n. 139, depositata in cancelleria il successivo 10 giugno. Nella seduta del 27 luglio 2016, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

dibattimentale penale. **Il Senato approva.** La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

rappresentante del Governo, senatrici e senatori, il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura è complesso e multiforme; coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri. È diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività. Gli ultimi episodi ci parlano, infatti, di intermediazione illecita e lavoro sfruttato in Toscana nella produzione del Chianti. Ci sono stati casi nel bresciano, sempre nella produzione di vini. In Emilia, oltre al fenomeno nella macellazione delle carni, sono stati segnalati casi nella raccolta delle pesche nettarine. Poi ci sono le situazioni estreme e molto conosciute come quelle della raccolta dei pomodori, degli ortaggi e della frutta nelle nostre Regioni del Sud. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono oggi inaccettabili e incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale. Il caporalato e lo sfruttamento del lavoro, in agricoltura come in altri settori, costituiscono un'aperta violazione degli articoli che tutelano i lavoratori nel Titolo III della Parte I della Costituzione italiana: mi riferisco agli articoli 36, 37 e 38. Le aziende e i datori di lavoro che si servono dell'intermediazione illecita dei caporali e sfruttano il lavoro di chi è in condizioni di bisogno, recano danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in primo luogo degli stessi lavoratori che sono costretti a condizioni di vita degradanti ed intollerabili. Inoltre, queste imprese svolgono la loro attività in palese contrasto con quell'utilità sociale che, secondo quanto sancito dall'articolo 41 della Costituzione, deve invece sempre caratterizzare l'iniziativa economica privata. altresì di ingiusti profitti costruiti sullo sfruttamento dei lavoratori, costringendo ad una concorrenza al ribasso le aziende e gli imprenditori onesti che assumono regolarmente, con conseguenze negative sul prezzo, sulla qualità e sulla stessa salubrità dei prodotti. Mi sembra interessante, a questo punto, rilevare che il fenomeno non è solo italiano. La Spagna, con la raccolta delle fragole nella provincia di Huelva, e la Francia in molti contesti rurali si confrontano anch'esse con il contrasto a simili fenomeni. Dicevo che è un fenomeno multiforme e presenta diverse strutture organizzative, a volte complesse, a volte molto semplici. I rapporti fra i soggetti in campo sono anch'essi molto differenziati e vanno da quotidiane relazioni di sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori per l'avvio a un lavoro caratterizzato da sfruttamento senza violenza e minaccia a, invece, situazioni in cui la violenza e la minaccia diventano esplicite. Un fenomeno del genere per essere affrontato ha bisogno di un intervento complesso che comprenda l'azione penale repressiva e la costruzione di politiche di prevenzione e contrasto. Infatti, questo intervento legislativo in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura si inserisce in un quadro di azioni messe in atto dal Governo relativamente a un incremento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Si tratta di un intervento essenziale. I dati delle ispezioni nel settore agricolo nell'anno 2015 ci dicono che sono state ispezionate 8.662 aziende per cento rispetto al 2014), sono stati individuati 6.153 lavoratori irregolari, 3.629 totalmente in nero, riscontrati 713 episodi di caporalato. Ci dicono che c'è piena regolarità solo nel 43 per cento dei casi, parziale irregolarità (lavoro grigio) nel 28,8 per cento, completa irregolarità (lavoro nero) nel 28 C'è stata poi l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro che accentra la vigilanza già esercitata dal personale INPS e INAIL, in modo da evitare controlli in sequenza dei diversi soggetti che influiscono sulla normale funzionalità delle imprese, ottimizzando risorse e rendendoli più efficaci.

con le parti sociali e le associazioni di volontariato. Il protocollo, che durerà fino a tutto il 2017, utilizza i fondi PON Legalità (Piani operativi nazionali, fondi europei per progetti sovraregionali) e FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) prova a rispondere alle situazioni più urgenti con interventi che vanno, tra gli altri, dalle convenzioni per il trasporto gratuito, all'istituzione dei presidi medico-sanitari, da progetti pilota di accoglienza per i lavoratori stagionali utilizzando temporaneamente immobili demaniali, alla sperimentazione di servizi itineranti con presenza di mediatori culturali. Inoltre, nel piano di intervento per le verifiche e i controlli ci si concentrerà nelle aree territoriali di maggiore vulnerabilità operando di concerto con il Ministero delle politiche agricole, con il Ministero dell'interno, utilizzando le competenze del Corpo forestale dello Stato e i dati sulle aziende agricole contenuti nelle banche dati di riferimento. Il protocollo interessa per ora cinque Regioni (tutte al Sud), individuate come a maggior rischio: è, comunque, un segnale chiaro a chi vuole operare nell'illegalità e speculare sullo stato di necessità di tanti lavoratori immigrati. Vengo adesso al merito del disegno di legge al nostro esame. Il disegno di legge governativo è stato presentato all'inizio del 2016. Per i primi cinque articoli interveniva con modifiche al codice penale e al codice di procedura penale relativamente a circostanza attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità legge conteneva poi, all'articolo 6, una serie di integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al decreto-legge n. 91 del 2014. Se negli articoli da 1 a 5 si configurava la parte repressiva del provvedimento, l'articolo 6 e il successivo articolo 7 fissavano le politiche di intervento per il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, in grado di affrontare l'urgenza e indirizzare le scelte di intervento future. Gli articoli 8 e 9 contenevano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Il 10 febbraio il provvedimento è stato incardinato in Commissione agricoltura

Come testo base è stato assunto il testo del Governo. Già dall'inizio della discussione in Commissione erano emerse con forza le difficoltà applicative del reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale; di particolare rilievo la comunicazione che in proposito ha fatto il ministro Orlando relativamente ai dati statistici relativi ai procedimenti per il reato di cui Il Ministro ha parlato di sole 34 iscrizioni presso gli uffici del gip e di otto procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale. Altro elemento problematico era la difficoltà, con l'attuale definizione di reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici di sfruttamento fossero riconducibili al datore medesimo, che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati. L'esperienza dei cinque anni dalla sua introduzione nel codice mostrano come l'attuale formulazione del 603-*bis* si sia dimostrata del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. A fronte di tali difficoltà, abbiamo deciso di riscrivere il reato in modo da renderlo applicabile e definendo al suo interno una figura di reato autonoma per il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, modulando le pene in relazione alla presenza di minaccia e violenza e rendendo meno rigidi e di più semplice valutazione gli indici di sfruttamento. L'inserimento di una figura autonoma di reato per il datore di lavoro si è riverberata chiaramente su tutti gli altri articoli del disegno di legge del Governo relativi alla parte penale. In particolare, l'inserimento della responsabilità diretta dell'impresa ha comportato l'applicazione di una serie di pene accessorie, che di fatto hanno raccolto molto dello sforzo emendativo che si è sviluppato nelle proposte presentate in Commissione, oltre a una serie di elementi presenti nel disegno congiunto a quello governativo. Penso sia il caso, a questo punto, di descrivere in modo dettagliato la riscrittura del reato e gli altri interventi sui primi cinque articoli del disegno di legge governativo assunto come testo base. Con l'articolo 1 si riscrive l'intero articolo 603-*bis* del codice penale, che, nella versione attuale, punisce nei fatti il solo caporale e richiede come requisiti del reato l'organizzazione di una attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. Si riscrive la condotta dell'intermediario e si punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore, che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minaccia. Si prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante l'uso di violenza o minaccia. Conseguentemente, si introduce una maggiore gradualità delle pene comprese quelle pecuniarie:

Si prevede la figura di reato autonoma del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, anche non avendola assunta mediante ricorso a un intermediario (da uno a sei anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, da cinque a otto con violenza o minaccia). Si precisano e semplificano gli indici di sfruttamento lavorativo, rendendoli più puntuali. In particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro, quando è reiterata e non solo sistematica come nel testo attuale. Dopo la riscrittura del reato, siamo intervenuti su una serie di modifiche al codice penale che il disegno di legge del Governo presentava. In particolare, al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa governativa abbiamo ridefinito l'attenuante. Per il ricorrere dell'attenuante si richiede ora che il responsabile, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. La più specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante è diretta conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro. Inoltre, viene aumentata la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante, dalla metà ai due terzi. La riduzione fino a due terzi è coerente con la diminuzione di pena prevista in relazione ad altre fattispecie incriminatrici e mira a rompere il sodalizio criminale che si instaura tra il caporale e il datore di lavoro, premiando quelle forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che permettono di estirpare il fenomeno. Nel testo oggi all'esame di quest'Assemblea si rinvia alle norme previste dall'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, che prevedono la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti. inoltre si esclude l'applicazione del 600-*septies*.1, per permettere l'applicazione dell'attenuante specifica di cui all'articolo 603-*bis*.l (e quindi anche della diminuente da un terzo a due terzi) anche ai concorrenti nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In relazione alla confisca obbligatoria inserita all'articolo 1 del disegno di legge del Governo e adesso contenuta all'articolo 2, abbiamo apportato le seguenti modifiche: che la suddetta faccia salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno e che la stessa previsione riguardi i beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona. Si introduce poi una nuova disposizione nel disegno 3, il controllo giudiziario dell'azienda disposto da parte del giudice, qualora ricorrano i presupposti indicati del sequestro preventivo, cui l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni gravi e negative sui livelli occupazionali, o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori giudiziari, che affiancano l'imprenditore nella gestione dell'azienda. Compiti dell'amministratore giudiziario saranno: il controllo del rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento; la regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'inizio del procedimento non erano regolarmente assunti; l'adozione di misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore. Viene poi introdotta, al quarto comma, una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto nei casi in cui è consentita la confisca e nei casi di confisca disposta ai sensi del nuovo 603-*bis*.2, nei quali si prevede l'applicazione del regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenute nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Infine si riformula la norma sull'arresto in flagranza, prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia. Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge del Governo, ora articoli 6 e 7, non sono stati oggetto di modifiche da parte della commissione referente, ma soprattutto sull'articolo 6, in tema di responsabilità degli enti, si riverberano gli effetti della riscrittura del reato. Il vecchio articolo 6 sviluppava, assieme all'articolo 7, la parte del provvedimento che fissava le politiche di contrasto al fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. All'articolo 6, adesso articolo 8, si interviene per modificare e arricchire la funzione e l'impatto della Rete del lavoro agricolo di qualità. Le integrazioni sono finalizzate a estendere l'ambito dei soggetti presenti sia nella cabina di regia che sovrintende al funzionamento della Rete, sia l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete. Entrano nella cabina di regia l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'ANPAL, l'Agenzia delle entrate. L'obiettivo di questi inserimenti è rendere più efficace l'intervento della cabina di regia soprattutto nella valutazione delle richieste di iscrizione e nella capacità di leggere a livello nazionale cosa succede nel settore agricolo nel nostro Paese e proporre interventi adeguati. Infatti, la cabina di regia procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo su base trimestrale anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, valutando in particolare il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato

Questo non comporterà modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli e contestualmente determina invece l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. Si adotta in questo modo il sistema di comunicazione mensile delle persone occupate attualmente vigente per le aziende non agricole, omogeneizzando i dati e i loro tempi di raccolta. Inoltre, nella cabina di regia si sono apportate modifiche e semplificazioni alle norme che definiscono i requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità. In particolare fra i requisiti è stata richiesta esplicitamente l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. L'obiettivo delle modifiche fatte è rendere più efficace l'intervento della Rete e più numerosa la platea degli aderenti confermando la volontarietà dell'adesione. A legislazione attuale si rilevano infatti molti problemi: ad ottobre 2015 erano appena 300, su un potenziale di 740.000, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Per quanto riguarda l'ampliamento dei soggetti che possono aderire alla Rete, si sottolinea la possibilità di aderire per gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i soggetti abilitati al trasporto delle persone e le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo Chiaramente i soggetti privati abilitati al trasporto di persone e quelli autorizzati all'intermediazione di manodopera possono aderire nel rispetto dei requisiti previsti per le imprese agricole. L'adesione di tali soggetti si concretizza con la creazione dei nodi locali della Rete presso le CISOA e il nodo diventa il punto più interessante per analizzare da vicino i problemi dell'agricoltura del territorio conoscendone livelli di meccanizzazione, specificità e difficoltà, per affrontare in modo sperimentale utilizzando buone pratiche, ad esempio gli elenchi di prenotazione, i due problemi principali che bisogna risolvere per contrastare il caporalato: il collocamento agricolo e il trasporto dei lavoratori sino al luogo di lavoro. Per quanto riguarda il collocamento, che dovrà basarsi sulla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, vanno attivate prima di tutto le conoscenze relativamente alla manodopera disponibile: quantità, capacità, qualità, specializzazione, esigenze del territorio, caratteristiche delle produzioni, ammodernamento dei sistemi produttivi. Poi, vanno impegnati tutti i soggetti in grado di fare intermediazione di manodopera in modo legale e trasparente e gli enti locali per fornire i supporti necessari. Per quanto riguarda il trasporto dei lavoratori, la norma prevede che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, rilasciata dalle autorità competenti, e in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione alla Rete, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Essi stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi. L'articolo 7 del disegno di legge governativo, ora articolo 9, affronta le urgenze che ogni anno, in specifici periodi si palesano in diversi territori. Infatti, prevede che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli, al fine di evitare i rischi legati al loro maggior afflusso. Il piano sarà oggetto di intesa con la Conferenza unificata e prevederà il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore. Il lavoro di Commissione ha aggiunto la necessità di idonee forme di collaborazioni con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Il provvedimento, nonostante non sia composto di molti articoli, è stato molto complesso: ha coinvolto tre Ministeri - politiche agricole, giustizia e lavoro - e io qui vorrei ringraziare i ministri Martina, Orlando e Poletti per l'impegno nel seguire il provvedimento. Ne è stata prova la loro presenza in Commissione con comunicazioni sul tema che sono state punti fondamentali del dibattito. Il provvedimento, poi, ha coinvolto in modo significativo oltre alla Commissione di merito anche le Commissioni lavoro e giustizia e giustizia e ringrazio la Commissione lavoro, in particolare la senatrice Parente, relatrice in Commissione, per l'articolato parere che ci ha offerto e per averlo illustrato in 9a Commissione. Allo stesso modo voglio ringraziare la Commissione giustizia tutta e in particolare il senatore Lumia, relatore del provvedimento. La Commissione giustizia mi ha ospitato in due delle sue riunioni in cui c'è stata una discussione approfondita sul testo che ha coinvolto tutti i Gruppi e il parere espresso ha segnato molto l'ultima versione del provvedimento. Devo poi dei ringraziamenti particolari ai membri della 9a Commissione, a partire dal Presidente, che con la discussione puntuale e la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno

La riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento è oggi fondamentale per una adeguata repressione del fenomeno e io, che non sono una giurista (si sarà capito), penso che la ridefinizione di questo riconduca il diritto penale alla sua principale funzione che è quella di rappresentare garanzie e tutele per chi è più debole. Per questo auspico che quest'Assemblea, dopo una adeguata trattazione, voti nel modo più allargato possibile il provvedimento e che la Camera lo tratti con l'urgenza necessaria. *(Applausi

Signor Presidente, come i colleghi hanno avuto modo di constatare, il lavoro svolto dalla Commissione agricoltura è stato preziosissimo e mette l'Assemblea nelle migliori condizioni per fare una scelta importante: fare in modo che nel nostro Paese sia finalmente combattuta con efficacia e con risolutezza la piaga del caporalato, la piaga dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Siamo noi della Commissione giustizia che ringraziamo la senatrice Gatti per il lavoro che ha svolto, per la tenacia, la cura

tutti d'accordo nel dire no al caporalato e poi nelle Aule del Parlamento si hanno atteggiamenti di freno, di disattenzione se non di boicottaggio delle varie iniziative che, in questi anni, si sono intraprese nelle Commissioni di merito. Finalmente siamo in Aula. Finalmente c'è una proposta equilibrata. Badate bene, colleghi, il mondo dell'agricoltura non ha paura del provvedimento esame, perché ha compreso sulla sua pelle che il rapporto tra legalità e sviluppo è una risorsa, non è una pietra d'inciampo, non limita le produzioni, non impedisce la possibilità di fare buoni profitti, non è un limite per espandere i nostri preziosissimi e qualificati prodotti nel mercato nazionale e mondiale. Certo, il caporalato non è più una piaga di alcuni territori:

Si è fatto un lavoro prezioso, che ci ha messo finalmente in piena sintonia con la tutela dei diritti umani, perché il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura degradano la dignità della persona, umiliano le sue caratteristiche, addirittura spesso riducono in schiavitù quel lavoratore, quella lavoratrice e quel bambino utilizzati nei campi.

Pensiamo al secondo e terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che disciplinano i limiti alla durata della giornata lavorativa, il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite, questioni lontanissime del tutto prive di qualunque prospettiva in una tale condizione di sfruttamento. Inoltre, non vi sono limiti di età, né tutele per le lavoratrici madri e solitamente le donne e i minori ricevono retribuzioni inferiori a parità di lavoro svolto caso in palese violazione degli articoli 37 e 38 della Costituzione, che richiamano alla sicurezza del lavoro, alla tutela in caso di infortunio o di malattia - e mai potranno godere di una pensione, come invece viene stabilito.

riscrive l'articolo 603-*bis* del codice penale, con cui finalmente si ridefinisce la condotta dell'intermediario e si punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga il lavoratore a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenze o minacce. Si prevedono delle aggravanti e anche delle interessanti attenuanti, perché l'obiettivo non è semplicemente punitivo, ma è anche quello di mettere nelle condizioni

In questo modo separiamo il destino del caporale, dello sfruttatore e mettiamo l'azienda agricola nelle condizioni di intraprendere un cammino, accompagnato, in alcuni casi, anche dagli istituti dell'amministrazione giudiziaria, per

con le decisioni della Commissione agricoltura, l'Assemblea è nelle condizioni di condividere il testo in esame, di farlo vivere nel nostro Paese e finalmente di dire in agricoltura legalità e sviluppo devono essere le uniche dinamiche in grado di far crescere il nostro prodotto e farlo diventare sempre più di eccellenza e di qualità anche sul versante dei diritti.

assolutamente descrittiva del processo e del risultato ottenuto in Commissione, nella quale ho rilevato un clima di particolare tensione collaborativa, volto proprio alla produzione di norme buone, ovviamente nel contemperamento degli interessi contrastanti. Vorrei fare una considerazione al riguardo. Della descrizione del lavoro dei campi, così duro e così aspro, e così aspro, è piena la letteratura dell'Ottocento, il Verismo, a volte con tratti oleografici, ma più spesso con momenti e pagine in cui è descritta con particolare asprezza la lotta per la vita dei braccianti, specialmente nelle campagne del Sud. Da allora a oggi sono successe due cose importanti. La prima è l'articolo 36 della nostra Costituzione, che ho già sentito citare, Costituzione che mette il lavoro come punto fondante della nostra Repubblica. All'articolo 36 - mi piace ricordarlo - è scritto che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». È scritto in modo articolato e preciso che il lavoro non è una merce.

al proprio sostentamento la partecipazione alla creazione di una società. Dopo questo passaggio, però, ce ne sono stati altri. è stata posta in essere una serie di attacchi e di resistenze di parti sociali che di questa Costituzione non sono amiche.

questo tipo di impostazione ha portato - ad esempio - alla pressione enorme che la grande distribuzione esercita sulle nostre imprese agricole, costringendole a margini di redditività estremamente bassi, al limite della sopravvivenza. sbagliando, una sorta di autogiustificazione per ritornare, dopo l'articolo 36 della Costituzione, a condizioni di lavoro che somigliano estremamente a quelle descritte dalla nostra letteratura dell'Ottocento. Ritornate, cioè, indietro nei secoli. Ritornare a uomini e donne che possono morire nei campi perché lavorano durante le ore meridiane sotto il sole, che "schiattano" mentre lavorano.

tant'è che è pressoché unanime la richiesta da parte degli operatori del settore e delle organizzazioni sindacali che il provvedimento sia approvato in Senato quantomeno prima della pausa estiva.

per cui dalla Commissione è uscito un testo che tutti noi commissari abbiamo votato.

da molti, è assai avanti. Ad avviso della Sinistra italiana, nella nostra tensione verso l'obiettivo, e cioè la riduzione fino all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, dobbiamo cercare una collaborazione tra tutti gli attori:

che assicuri il consumatore del fatto che un dato prodotto non è frutto di sfruttamento.

appesantimenti ideologici. L'ultima ideologia rimasta, tanto forte da essere assurta al rango di verità, è l'attaccamento di tanta parte della nostra politica al mercato. Il mercato privato non risolve tutto; il mercato, anzi, può e spesso crea problemi. Per alcuni versi, l'intervento di un pubblico efficace ed efficiente può avere un ruolo importante.

cento. Mi chiedo: se queste somme fossero destinate al potenziamento degli uffici di collocamento e al loro funzionamento ottimale, efficace ed efficiente, non saremmo tutti più tranquilli? Non saremmo tutti più tranquilli se fosse lo Stato a svolgere la necessaria opera di intermediazione per reclutare quelle braccia che vanno a raccogliere sui campi?

esame è un provvedimento che il mondo dell'agricoltura attende da parecchio tempo e su cui si è lavorato in Commissione in maniera decisamente proficua e anche importante. Dico questo per richiedere attenzione al Ministro, che - finalmente - vedo presente in Aula,

Signor Ministro, che cosa è accaduto qualche ora fa in Commissione? Sottolineo che questo è accaduto non qualche settimana fa, ma poche ora fa. Improvvisamente è arrivata una velina, con un indirizzo politico

improvvisamente ci siamo trovati con una seduta convocata non dall'oggi a domani, ma dal pomeriggio per la sera, e con una votazione che ha falciato tutti gli emendamenti di opposizione. Forse uno o due ordini del giorno sono stati emendamenti che nascevano - come era noto anche al Governo - dal confronto con le associazioni di categoria del settore agricolo

Abbiamo dichiarato che non ci saremmo opposti a questo provvedimento, ritenendolo importante, ma certamente il metodo utilizzato dal Governo è pari al fenomeno che il provvedimento affronta: un metodo da caporali. Signor Ministro, non ci è sfuggito che lei, il giorno dopo, ha rilasciato delle dichiarazioni che leggo testualmente: «La Commissione agricoltura del Senato ha concluso i suoi lavori sul disegno di legge caporalato. Soddisfatto il ministro Martina: molto bene l'approvazione di oggi in Commissione agricoltura al Senato della nostra proposta di legge contro il caporalato. Ora servono sforzi in più. Approviamola in Aula entro luglio». Che sia una vostra proposta di legge è scritto sul testo,

di andare, ancora una volta, a chiedere a chi rispetta già le leggi - cioè gli onesti - di rispettarne di ancora più severe, trascurando il fatto che i disonesti, per definizione, le leggi non le rispettano. E porto un esempio molto semplice. Noi importiamo

di tutela e di rispetto del lavoro in agricoltura. Su questi prodotti in questo provvedimento il Governo non si inserisce alcunché. Noi continueremo a importare i pomodori dal Nord Africa, piuttosto che da altri Paesi, o il riso, che viene dall'Oriente: prodotti dell'agricoltura che vanno sul nostro mercato, prodotti che nascono dallo sfruttamento della manodopera. Se un reato come questo deve esistere, deve essere universale. Sul nostro mercato e su quello europeo non deve esserci alcunché prodotto sfruttando la manodopera, come fa il caporalato. Altrimenti, avremo illuso un'altra volta il

Ancora una volta, altrimenti, resta la delusione di vedere un Governo e un Ministro che pensano di più a lavorare per fare apparire una certa immagine, che invece è molto lontana dalla concretezza di cui ci sarebbe bisogno.

strumento lo applicate solo a ciò che vi interessa, perché la narrazione data al Paese parla di un Parlamento che non sa lavorare e di un Governo molto efficiente che interviene con determinazione. Non abbiamo bisogno di queste dimostrazioni di retorica. Lei adesso sarà libero di fare la sua replica e di dire che tutto ciò è fuori da ogni fondamento. Lo vedremo nei prossimi giorni. Io rilancio una proposta avanzata in Commissione; faccia una breve riunione tra i Capigruppo; si definiscano punti di contatto e di sintesi tra le proposte giunte dal mondo agricolo, da Agrinsieme, su questo provvedimento;

La collega Gatti e tutti noi ci abbiamo messo una grande passione e tutti avevamo una forte urgenza di portarlo a termine. Questo vogliamo ribadire e lo vogliamo prima della raccolta. Non si raccontino altre fiabe, altre storie, altri film. Sarà il suo film, caro collega Candiani, ma non è la realtà.

turbano il nostro Paese. Si verificano in più di un comparto, specialmente nell'agricoltura e, in particolare, con riferimento alla raccolta agricola, dove la frequenza è massima. Le organizzazioni agricole più volte hanno evidenziato anche nelle audizioni - ne ho sentite molte, senatore Candiani - che la presenza del lavoro nero e del caporalato in agricoltura costituiscono un gravissimo

Esse si trovano a competere con le aziende del sommerso, che operano nell'inadempienza, con conseguenti costi di produzione nettamente inferiori. Il fenomeno incide sui lavoratori dipendenti, spesso privi di copertura previdenziale e assistenziale - lo ha ben detto in tutti i suoi passaggi la senatrice Gatti privi di un'idonea tutela sul piano della sicurezza. E non si può sottacere che la questione in alcuni territori e contesti economico-sociali sia di ordine pubblico. Le imprese non sono immuni dal rischio

dal Nord-Est. La Fincantieri, nel territorio da cui provengo, ha visto più volte impiegate le Forze dell'ordine e la magistratura. Processi e condanne inducono ad approfondire il tema e a inquadrare un ambiente in cui il reclutamento dei lavoratori avviene in un contesto non sempre estraneo

di un disegno di legge condiviso - lo sottolineo - da molte parti, dalla stragrande maggioranza di noi. Individua strumenti di contrasto per far fronte a un diffuso e dilagante problema. Sono circa 1.200.000 i lavoratori del comparto agricolo in Italia, di cui il 42 per cento in nero. Le agromafie muovono un giro di affari che, secondo i dati ISTAT e FLAI CGIL, tocca vertiginosamente i 2,5 miliardi di euro. Il caporalato è parte è parte di questo preoccupante sistema. Eccome se era urgente! È interessante e confortante che il rafforzamento dell'attività di verifica abbia portato da circa 5.400 accertamenti nel 2014 a 8.600 nel 2015.

di cui 3.600 in nero e circa 180 extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Il tasso di irregolarità ha riguardato oltre la metà delle verifiche.

Dal ciclo di audizioni della Commissione è emersa con chiarezza la necessità di intervenire sul reato di cui all'articolo 603-*bis*, più volte richiamato in questa sede, sanzionando i caporali, i datori di lavoro e le imprese che si avvalgono di tale metodo, modulando le responsabilità e riscrivendo il reato. Il caporalato può sostanziarsi in una serie articolata di operazioni, per cui occorre intervenire con una molteplicità di strumenti di contrasto. È fondamentale il versante non soltanto della

si prevede la pubblicazione di elenchi di aziende virtuose che volontariamente si iscrivono alle Rete. Le imprese ammesse alla Rete compaiono in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet dell'INPS - lo ha in precedenza citato la relatrice Gatti - e non sono ricomprese negli orientamenti dell'attività di vigilanza adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'istituto previdenziale, che devono invece concentrare i controlli sulle aziende non iscritte alla Rete. La Rete, così come è prevista attualmente, favorirebbe l'auspicata *intelligence* nell'attività di vigilanza. Quindi, il costante monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, le iniziative sull'organizzazione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori immigrati sono misure, oltre che di contrasto, di civiltà. La Rete di qualità costituisce, dunque, un importante impegno e una scelta innovativa per favorire un corretto andamento dell'attività delle imprese: essa dovrebbe intervenire anche con modalità sperimentali nel campo dell'intermediazione del lavoro agricolo, attraverso un approccio integrato, ad esempio con le commissioni provinciali per l'integrazione quindi importante la collaborazione con gli enti locali: un passaggio ritenuto necessario per vari aspetti che interessano il fenomeno del caporalato, tra cui il trasporto nelle zone agricole.

potenziata anche attraverso una maggiore diffusione sul territorio delle buone pratiche, soprattutto attraverso una forte e veloce sburocratizzazione. Anche questo è stato un lavoro e un impegno molto forte L'impegno è dunque concentrato sia sulla repressione delle condotte illecite, che tutelerà e farà crescere il fatturato delle imprese agricole che agiscono nella piena legalità, che - come ho detto - sulla prevenzione.

Non deve verificarsi più quanto accaduto ad Andria, fatto che abbiamo esaminato nella Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro: mi riferisco al decesso della lavoratrice agricola signora Paola Clemente. È emerso in Commissione di inchiesta, anche in quell'occasione, un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari:

di maggioranza che di opposizione, che hanno dato veramente il massimo e hanno consentito di arrivare alla condivisione larga di un provvedimento che rappresenta un passo in avanti di civiltà per il nostro Paese e per un lavoro agricolo di qualità.

Il tema potrebbe essere il seguente: perché arriviamo alla fine dell'estate con questo provvedimento?

nero. Si sta facendo, però un lavoro straordinario. Stiamo tentando di arginare un odioso fenomeno, che è fonte di infiltrazione, di tutto e di più, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Lo ha affermato vibratamente anche la relatrice, che ringrazio per il lavoro svolto,

fare qualche considerazione perché il provvedimento si potrebbe anche ascrivere a un sistema sanzionatorio: che cosa stiamo facendo con questo provvedimento? Sanzionare di più. Per evitare di sanzionare di più dobbiamo mettere le imprese agricole

controlli, una storia ampiamente segnalata non solo da me, ma da tanti colleghi. Ho apprezzato molto una norma attribuita a lei, signor Ministro, volta a sintetizzare i controlli su un organismo. Per quanto mi risulta, signor Ministro, ancora c'è la vecchia procedura: un'impresa agricola

questioni formali. Questo è un fenomeno che capita ormai da lunghissimo tempo, non lo stiamo scoprendo adesso: stiamo parlando da decenni di questa situazione. Invece bisogna colpire seriamente le aziende per le quali è nato questo provvedimento. Bisogna saper individuare

controllare. Signor Ministro, spero che questo provvedimento possa davvero correre e avere immediata attuazione e che possa traguardare a un minimo di risultato, quello di fare, come stiamo facendo, una battaglia di civiltà. Io e il mio Gruppo ci crediamo e avremo modo, in corso di dichiarazione di voto, di esprimerci favorevolmente sul disegno di

per sterile polemica, ma perché se è un'accusa ricorrente, è quella di usare troppo spesso la decretazione d'urgenza rispetto ai temi e alle problematiche che ci troviamo ad affrontare. In questo caso, il Governo ha tempestivamente percorso la strada opposta, cioè quella del coinvolgimento parlamentare e quindi di tutte le forze politiche, proprio su un provvedimento che in questi anni non solo ha fatto parlare tanto l'opinione pubblica ma di certo non qualifica il nostro Paese ed il lavoro: in questo caso non ha qualificato

Fasiolo, intervengo come Presidente della Commissione d'inchiesta per gli infortuni sul lavoro che ha dedicato una parte importante del suo impegno al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in questo caso partendo da alcuni fatti, anche molto tristi, della cronaca del nostro Paese, a partire dal decesso della signora Paola Clemente - lo ricordo ai colleghi all'Assemblea del Senato

La Commissione non si limitò ad analizzare il decesso della signora Paola Clemente, svolgendo un ciclo di audizioni molto compiuto, ma provò, da quella esperienza, anche a tracciare un elenco delle questioni

sono alla base della volontà non solo del Governo ma di questo Parlamento e sicuramente del Partito Democratico di intervenire su un tema che squalifica, come dicevamo, non solo il lavoro agricolo nel nostro Paese

emersero da quell'indagine. Riferisco, per dovere di cronaca, che il lavoro della nostra Commissione non finì con l'indagine sulla signora Paola Clemente, perché poco più di due mesi fa la stessa Commissione si è recata, con un'ispezione vera e propria, in un'azienda dell'agro pontino nella quale sono impiegati oltre 100 lavoratori indiani, sempre allo scopo di verificare se sussistano condizioni di caporalato nel settore agricolo, non solo evidentemente in Puglia, ma in varie parti del nostro Paese. La situazione che abbiamo trovato, e per la quale stiamo ancora finendo il nostro lavoro di approfondimento e di indagine, è legata ad alcuni dei temi che - lo ripeto - sono contenuti nel presente disegno di legge.

a quello del lavoro sommerso. Il disegno di legge che, come è stato ben ricordato, modifica l'articolo 603-*bis* del codice penale, interviene su alcune delle che abbiamo proposto come Commissione d'inchiesta e che sono state oggetto di emendamenti che abbiamo presentato e di ordini del giorno approvati. Tra le novità introdotte vi sono la confisca obbligatoria e l'arresto in flagranza di reato, la responsabilità amministrativa a carico dell'ente dell'ente privato, l'utilizzo dei proventi delle confische (ovviamente in questo caso inerenti al delitto in esame) assegnati al Fondo per le misure anti-tratta, la modifica della possibilità di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Viene specificato bene che tale adesione non è obbligatoria,

e civiltà, perché ritrovarsi a indagare su fatti che non si può immaginare che ancora esistano nel nostro Paese impone un'accelerazione e una condivisione anche nella scelta. Ritengo importante quello che si è fatto

mesi. Auspicheremo alcune altre modifiche, di cui ragioneremo anche più avanti, quali un più puntuale coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL, un più puntuale raccordo delle Forze dell'ordine impegnate in tema

non vada bene. Probabilmente se non fosse stato così, anche le condizioni della signora sarebbero state verificate molto prima. È questo uno dei temi sui quali ci sentiamo impegnati e sui quali vogliamo continuare a lavorare insieme al Governo

Signora Presidente, colleghi senatori, siamo qui in Aula oggi, in questo afoso mese di luglio, per affrontare la discussione relativa a un disegno di legge che a me, come a tanti di noi, sta sta particolarmente a cuore. Il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, di cui discutiamo, è di fondamentale importanza poiché il tema non è più rinviabile. L'estate del 2015 è passata alla storia come quella che ha comportato nelle nostre campagne il bilancio più pesante in termini di perdita di vite umane. Quello del caporalato è un fenomeno drammatico e purtroppo antico, ma negli ultimi decenni ha assunto caratteristiche nuove, in quanto molti braccianti e molti caporali sono di origine non italiana. Le cronache riportano spesso episodi tragici nei campi di pomodori della Puglia. Non dimentichiamoci però che il caporalato non è un fenomeno endemico del Sud Italia, ma coinvolge molte altre Regioni: dalla Lombardia al Veneto, dall'Emilia-Romagna alla Toscana, tutta l'Italia deve fare i conti con la condizione drammatica in cui vivono e lavorano decine di migliaia di lavoratori italiani e stranieri nelle nostre campagne. In cuor mio penso che nel 2016 non sia in alcun modo accettabile che nel nostro Paese ancora si muoia di lavoro, di fatica, di caldo nei campi, che siano di pomodori, arance o vigneti. Non è giusto, non lo è in nessuna epoca, tantomeno può esserlo al giorno d'oggi. Eppure, purtroppo, è ancora così. C'è ancora chi muore di lavoro, e che sia straniero o italiano, uomo o donna non è affatto rilevante. Secondo indagini recenti l'anno scorso le vittime del caporalato sarebbero state almeno dieci, ma tra i quattrocentomila braccianti agricoli in Italia, sono oltre centomila i lavoratori che si trovano in condizioni di lavoro di paraschiavismo e quarantamila quelli a rischio di sfruttamento. Di questi, il 60 per cento lavora senza avere accesso a servizi igienici o all'acqua corrente cento si ammala di malattie legate allo sfruttamento. Tutto questo per una cifra che va, nel migliore dei casi, dai 25 ai 30 euro al giorno, per turni da dieci, dodici ore consecutive. Sto riportando quanto asserito in uno studio basato sui dati della Federazione lavoratori agroindustria della CGIL, la quale segnala che i lavoratori sfruttati dal caporalato, nell'80 per cento dei casi sono stranieri, come ben sappiamo arrivati in Italia in cerca di fortuna e costretti in condizione di schiavitù a lavorare nei campi per pochi euro l'ora. I dati dello studio denunciano condizioni di lavoro indecenti in decine di casi. Inoltre, il caporalato sottrae alle casse dello Stato circa 600 milioni di euro all'anno, mentre i lavoratori sfruttati guadagnano meno della metà rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale. Con i soldi guadagnati, poi, i lavoratori non sono in grado di garantirsi un'esistenza dignitosa, né di acquistare i medicinali necessari per curare la propria salute, visto che chi svolge lavori pesanti nei campi per più di dodici ore al giorno in ogni condizione climatica è ovviamente esposto a ogni tipo di malattia e infortunio, malattie che peraltro sarebbero curabili con comunissimi farmaci ma, se manca il denaro per acquistarli, i disturbi vengono tralasciati e diventano cronici. Purtroppo, la pressione migratoria che investe il nostro Paese negli ultimi anni, in combinazione con la crisi economica, spinge e incoraggia imprenditori senza scrupoli a ridurre i costi di produzione attraverso lo sfruttamento della manodopera a basso costo, trasformando interi settori produttivi e danneggiando le migliaia di imprese sane e oneste che vengono sopraffatte da questa infame forma di concorrenza sleale. In questo contesto, è la criminalità organizzata a trarre i maggiori profitti, dando vita al fenomeno detto delle agromafie, pronte a sfruttare la vulnerabilità dei lavoratori migranti e la condizione di difficoltà di tanti lavoratori italiani rimasti disoccupati. Secondo i dati del secondo rapporto «Agromafie e Capolarato» dell'Osservatorio Placido Rizzotto, il caporalato controlla un giro di affari miliardario, diffuso in tutta Italia. Non dobbiamo dimenticare, poi, il ruolo delle multinazionali del settore della trasformazione agricola, che con l'imposizione di prezzi di acquisto sempre più bassi, costringono le aziende agricole a produrre sottocosto, a chiudere, oppure, nel peggiore dei casi, a ricercare metodi illeciti per abbattere i costi di produzione. L'introduzione di modifiche legislative, volte a garantire una più efficace azione di contrasto del fenomeno, è sicuramente un passo necessario e importante, e per questo impegno ringrazio il Governo e in particolare i ministri Martina, Poletti ed Orlando. Come ho avuto più volte occasione di ripetere, avendo peraltro l'onore di fare parte della Commissione antimafia, bisogna partire dalla repressione dell'illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori, in violazione delle più elementari norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei diritti fondamentali della persona, perché è di un vero e proprio fenomeno mafioso e criminale che stiamo parlando. Le modifiche al codice penale che prevedono un inasprimento degli strumenti a disposizione della magistratura e delle Forze dell'ordine non possono che essere condivise, sia nel caso dell'estensione dell'arresto obbligatorio e della confisca obbligatoria al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sia nel caso dell'introduzione di una circostanza attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e per assicurare le prove dei reati e l'individuazione degli altri responsabili, in modo da squarciare il velo di omertà di cui troppe volte ci siamo tristemente occupati. Altrettanto lodevole è la previsione di un fondo per indennizzi alle vittime del delitto di caporalato, equiparate alle vittime di tratta, così come l'introduzione di un piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali. La lotta alle mafie deve essere la stella polare dell'azione del Governo e del Parlamento. Il danno economico e sociale causato dalla criminalità organizzata deve essere ridotto al minimo, al fine di recuperare quante più risorse possibili da destinare all'economia sana e virtuosa di questo nostro amato Paese. Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura in particolare, accanto a un sistema di misure che puniscano le imprese che si rendono complici dello sfruttamento illecito della manodopera, dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi al fine di

e che non approfittano dei lavoratori al fine di realizzare profitti illeciti. Bisogna introdurre un severo controllo della filiera produttiva, con verifiche in ogni fase della produzione, dalla raccolta alla trasformazione industriale sino alla vendita al dettaglio. Solo garantendo agli imprenditori onesti un giusto ritorno per i loro sforzi, saremo in grado di eliminare i vantaggi che si ottengono utilizzando forme di lavoro illegali. Per questo motivo, plaudo anche all'introduzione della certificazione etica del lavoro agricolo e alla costituzione di una cabina di regia che metta insieme INPS, sindacati, organizzazioni agricole e istituzioni. Anche il *report* dell'ISTAT sulla struttura delle aziende agricole, pubblicato lo scorso settembre, conferma l'importanza del lavoro agricolo di qualità e del valore

I dati di vendita ci dicono che i consumatori sono disposti a premiare le aziende che possano certificare sulle loro confezioni il rispetto di determinati *standard* qualitativi. Penso, ovviamente, alle certificazioni delle produzioni biologiche e organiche, ma il ragionamento si potrebbe tranquillamente estendere a una certificazione che garantisca il rispetto dei più elementari diritti dei lavoratori. E allora ben venga la Rete del lavoro agricolo di qualità e le articolazioni territoriali della sua cabina di regia. Concludo rivolgendo un pensiero alle vittime del lavoro nei campi e alle loro famiglie. Sono soprattutto le donne che prestano il loro corpo a questo duro lavoro e che hanno offerto il più pesante tributo: la loro stessa vita. E allora il mio pensiero va, una tra tutte, a Paola Clemente, già ricordata più volte in Assemblea oggi: 49 anni, morta di infarto nelle campagne di Andria. Un triste destino che non può essere accettato nella nostra società che vuole essere all'avanguardia nella protezione dei lavoratori e dei loro diritti. Procediamo, dunque, onorevoli colleghi senatori, con l'approvazione di questo disegno di legge, affinché il dramma delle morti nei campi di tutta Italia sparisca dalle cronache dei giornali e resti solo un triste ricordo di un passato che ci siamo lasciati alle spalle.

condivido la relazione della collega Gatti sulla necessità e, in qualche modo, l'urgenza di una legge per contrastare il caporalato, che alcuni giustamente definiscono una piaga. Ciò è vero, soprattutto in alcuni territori dove a causa del caporalato l'organizzazione del lavoro passa

ma soprattutto a Rignano, con la raccolta del pomodoro, dove sorge un ghetto che racchiude i migranti e che è stato oggetto di tante inchieste giornalistiche a livello internazionale, proprio per la disumanità delle condizioni di vita. Si tratta di un ghetto che, nonostante l'impegno della Regione Puglia e l'interessamento anche del Viminale, è purtroppo ancora lì, a riprova di un fenomeno per cui non sono sufficienti solo misure repressive, ma che ha un suo radicamento sociale in cui il caporale svolge una funzione centrale per il mantenimento di quell'odioso sistema, come provato dalle audizioni che abbiamo svolto in Commissione.

le produzioni non riescono o non intendono fare sistema, creare consorzi, aumentare il proprio valore complessivo, anche agli occhi della trasformazione e della distribuzione, e che fa leva ancora sull'abbattimento del costo del lavoro. Per questa ragione credo che il contrasto al caporalato passi anche dalla capacità di ammodernamento di sistemi e ambiti produttivi che sono rimasti clamorosamente indietro che non riescono essi stessi ad attribuire il giusto valore al loro prodotto: si tratta di un aspetto da non sottovalutare anche rispetto alla proposta che stiamo discutendo e in cui vi sono altresì responsabilità da parte dell'ente pubblico. Dobbiamo essere molto bravi a costruire norme che tengano conto del fatto che il fenomeno si circoscrive in determinate aree per combatterlo meglio, ma anche per non far ricadere su quei sistemi produttivi in cui fenomeno è assente (il territorio da cui provengo è uno di questi) tutta una serie di norme e regole che, in prospettiva, potrebbero produrre un semplice inasprimento burocratico a fronte di un problema che, nei fatti, non esiste. esiste. Anche i colleghi della Commissione agricoltura sanno quante volte ho rilevato come il settore agricolo sia oberato da molta, troppa burocrazia. La nostra perplessità, già espressa con riferimento a precedenti provvedimenti normativi, sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, piuttosto che sulla cabina di regia è nota.

Abbiamo presentato molti emendamenti in Commissione. Alcuni sono stati accolti, altri assorbiti all'interno degli emendamenti della relatrice, altri sono stati respinti. Ringrazio, in particolare, la la relatrice Gatti, che sull'articolo 6 ha svolto un lavoro di grande mediazione ed è stata disponibile a rivedere l'intero articolo ed anche ad ammorbidirlo, per certi versi, rendendolo, per quanto ci riguarda, più facilmente applicabile. Sono anche soddisfatto che sia stato rimosso il riferimento all'indice di congruità occupazionale che rischiava di penalizzare proprio le aziende efficienti, quelle che sapevano ottimizzare l'uso

che il periodo di raccolta varia a seconda delle condizioni climatiche e che vi sono motivi che a volte impongono l'anticipo o il posticipo della vendemmia o della raccolta. Quindi, è un settore nel quale è difficile fare previsioni precise e l'introduzione di un sistema Uniemens in maniera precisa come per gli altri settori sarebbe stato un problema e sono naturalmente soddisfatto che sia stato accolto il nostro emendamento, con cui sono stati prorogati i termini di introduzione

vorrà accettare, con cui precisiamo che comunque rimane fermo l'obbligo del versamento trimestrale dei contributi agricoli unificati, per non imporre anticipazioni che possono creare qualche problema alle aziende. Abbiamo presentato in Aula anche altri emendamenti, in particolare uno, firmato insieme al collega Berger, sulla possibilità,

le regole sono rispettate e dove le aziende sono abituate a rispettare le norme, questa potrebbe essere una semplificazione burocratica importante e interessante. Invito quindi il Governo a tenere anche se in sede di primo esame in Commissione è stato respinto. Abbiamo presentato in Aula anche alcuni emendamenti per ridurre gli effetti penali di alcuni

che prevedono che, in caso di errori fatti in buona fede o non importanti, si possa distinguere tra l'illecito grave e un illecito più lieve. Sono emendamenti assolutamente puntuali puntuali che chiedo al Governo di poter esaminare anche nei particolari, sperando che almeno qualcuno possa essere accolto. Abbiamo presentato anche un emendamento per chiarire meglio la posizione delle cooperative agricole che forniscono servizi nel sistema trentino e altoatesino come sapete, più del 90 per cento della produzione agricola è organizzata in cooperative, che a volte forniscono anche servizi per il trasporto, l'alloggio e le regolarizzazioni. Questo, naturalmente, non è caporalato ma fornitura di servizi che è perfettamente regolare, ma l'emendamento lo avrebbe precisato

quei servizi che sembrano rendere indispensabile l'utilizzo del caporalato. Sono proprio gli enti locali o, comunque, le cooperative di lavoro, le realtà che si occupano del territorio e che possono sostituire il caporalato nell'organizzazione di servizi che siano giusti, regolari e, soprattutto, rispettosi dei diritti dei lavoratori.

cercare di non vanificare l'efficacia di un testo che vuole arrivare non dico in maniera definitiva, ma quantomeno incisiva al cuore del problema e iniziare a risolverlo cercando però di tener conto di chi non ha nulla a che fare con il

particolare e per questo non posso che ringraziare tutta la Commissione, la relatrice Gatti e il vice ministro Olivero, assieme a tutti i colleghi, perché ha seguito direttamente e in maniera molto precisa

Grazie, Presidente.

ogni qualvolta le attività stagionali richiedono un uso di manodopera superiore alle necessità medie che si manifestano nel corso dell'anno. Si tratta di una vera e propria economia sommersa che genera enormi profitti, distorce la concorrenza e alimenta una malavita particolarmente violenta che controlla oltre 300.000 persone. Le indagini delle Forze di polizia e anche quelle giornalistiche ci hanno indicato che i settori più esposti al caporalato sono l'agricoltura e l'edilizia, ma anche quello manifatturiero e turistico. I soggetti che subiscono di più lo sfruttamento sono gli extracomunitari, in particolare quelli senza permesso di soggiorno. In questo contesto non mancano neanche immigrati che si trasformano da vittime in sfruttatori di altri immigrati o realizzano complicità con le organizzazioni criminali. Il testo che licenzieremo prevede migliori tutele per i lavoratori e identifica pene mirate e graduate per coloro che mettono in pratica il reato di caporalato. Il tutto è stato possibile attraverso un lavoro certosino della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, che ha operato profonde e significative modifiche al testo originario licenziato dal Governo; un lavoro che ha visto maggioranza e opposizione lavorare alacremente e insieme per un quadro giuridico che fosse il più compiuto possibile. Oltre alla parte penale e sanzionatoria, il disegno di legge contiene una parte relativa alle politiche di prevenzione e contrasto al fenomeno, con la Rete del lavoro agricolo di qualità. La Rete, attualmente costituita solo dalla cabina di regia, si articola nel territorio coinvolgendo tutti i soggetti in grado di affrontare i due problemi del caporalato: l'organizzazione del collocamento agricolo e quella del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro. Si tratta di un passo importante, che prova ad affrontare un problema, che segna negativamente non solo l'agricoltura, ma anche altri settori, e mette a rischio la qualità dei nostri prodotti. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono inaccettabili e incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale. Questo provvedimento è atteso da molto dalle parti sociali e da tutto il Paese, e ci auguriamo che possa essere approvato con il più largo consenso. Per quanto riguarda gli aspetti penali, in Commissione Commissione si è riscritto l'intero articolo 603-*bis* del codice penale, che oggi punisce solo il caporale e richiede, come requisiti del reato, l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. L'esperienza dei cinque anni dalla sua introduzione nel codice mostra come l'attuale formulazione dell'articolo 603-*bis* sia del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. La nuova formulazione riscrive la condotta dell'intermediario e punisce anche quella singola del datore di lavoro o utilizzatore, che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minacce. Nel caso in cui vi sia uso di violenza o minaccia, è prevista un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento: infatti, se è stabilita la reclusione da uno a sei anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, con la presenza delle stesse la pena va da cinque a otto anni. Si precisano e si semplificano, inoltre, gli indici di sfruttamento lavorativo, rendendoli più puntuali: in particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro quando è reiterata e non solo sistematica, nonché la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Aggravanti specifiche, che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà, sono il reclutamento del numero di lavoratori superiore a tre, la minore età dei lavoratori reclutati e l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo. L'articolo 2 prevede invece delle attenuanti nei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, se il responsabile dimostra di cooperare, ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. l'obbligatorietà della confisca delle cose servite o destinate a commettere il reato, fatti salvi, in ogni caso, i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. Si possono confiscare le cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, i beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto. Altra novità rilevante introdotta in Commissione è la previsione nei procedimenti penali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, della possibilità da parte del giudice di disporre il controllo giudiziario dell'azienda, qualora ricorrano i presupposti indicati del sequestro preventivo, al fine di non creare delle ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. I reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commessi con violenza o minaccia vengono finalmente inclusi tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio, nei casi in cui gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato. Come esposto, notevoli sono i punti di rilievo di questo provvedimento. Mi preme ringraziare il presidente della Commissione, la Commissione stessa e soprattutto la relatrice Gatti, per la professionalità e la cooperazione avuta in Commissione. Il voto su questo provvedimento rappresenta un netto contrasto a una patologia del sistema, che crea economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri di mercato. Si cerca di combattere in modo definitivo la criminalità italiana e straniera, che si avvale di manodopera irregolare o in nero, riducendola in schiavitù, violando i diritti umani, falsando gli equilibri di mercato e recando danno anche alle nostre imprese, che invece operano nella regolarità. Questo significa lavorare per per garantire la sicurezza del Paese. Pertanto, auspico da parte dell'Assemblea un voto unanime: sarebbe una bella pagina per l'agricoltura e una bella pagina per il Paese.

modificando la legislazione vigente, consentiranno di punire in maniera robusta e di inquadrare in maniera più veloce ed efficace i casi di intermediazione illecita della manodopera nel settore dell'agricoltura. Il provvedimento inserisce delle fattispecie sanzionatorie nuove, che ci vedono, come Movimento 5 Stelle, assolutamente unanimi nel ritenere che siano positive. Certo è che c'è una parte su cui la Commissione giustizia aveva espresso un parere alla Commissione agricoltura, chiedendo che alcune pene fossero

si vanno a introdurre delle norme che vogliono proprio debellare questo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo.

quando si vanno a infliggere le sanzioni per coloro che sfruttano, in maniera amorale,

voluto anche irrobustire le pene in riferimento alla confisca dei beni. In particolare, volevamo che si inserissero delle norme che andassero a confiscare le cose impiegate o destinate a commettere reato, reato, le cose senza prezzo (quindi il prodotto o il profitto), nonché il ramo d'azienda, commerciale o agricola, ovvero il fondo rustico impiegati o destinati a commettere reato.

era importante, anche come strumento che evitasse giochetti e che, in un certo qual senso, dicesse a questi malfattori: non ti permettere di sfruttare un altro essere umano, perché altrimenti la pena che ti vado a comminare è veramente forte e ti tolgo anche i beni che ti sono serviti per commettere quel reato.

delle proposte che non hanno dietro assolutamente nessun tipo di bandiera ideologica: sono delle proposte di buonsenso che si fondano anche -

i controlli e offrire agli enti preposti al controllo degli strumenti molto più efficaci, in particolare, andando a ottimizzare gli indici di congruità occupazionale,

dobbiamo anche riconoscere che oggi, a far data dall'anno 2014, è stata istituita la cosiddetta Rete del lavoro agricolo di qualità. fa assumere a questo nuovo istituto una connotazione abbastanza importante. Prima ascoltavo un collega che ha affermato che forse era meglio inserire un altro strumento che potesse realmente dare un'indicazione più precisa all'organizzazione del lavoro agricolo di alcune aziende, in modo tale che il consumatore fosse consapevole che, con quel bollino, in un certo qual senso quel prodotto avesse un certo

un'ancor più importante connotazione all'interno del controllo che il consumatore può effettuare sul prodotto. Perché Perché è importante inquadrare bene oggi cos'è la Rete del lavoro agricolo di qualità? Perché in realtà con l'introduzione di queste norme capiremo se il soggetto che ha prodotto quel bene sta rispettando delle norme minime. Questo

Noi però riteniamo che si debba fare di più per migliorare questo importante istituto che è la Rete del lavoro agricolo di qualità. Pertanto, abbiamo offerto i nostri emendamenti che migliorano e cancellano anche quelle posizioni che potrebbero favorire alcune aziende. I nostri emendamenti fanno in modo che chi sta all'interno di questa Rete e chi sta all'interno della regia non sia in una posizione che lo possa favorire. Quindi noi speriamo che realmente il Governo, e quindi anche la maggioranza, si renda conto che c'è questa Rete agricola del lavoro di qualità che assume un ruolo molto importante e bisogna fare in modo che le persone che ci sono dentro non abbiano poi un tornaconto personale nel momento in cui assumono questi incarichi. PRESIDENTE.

e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Anche la Commissione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui faccio parte, si sta occupando ormai da mesi - lo ha ribadito poco fa nel suo intervento la presidente Fabbri attraverso sopralluoghi e audizioni, di questo preoccupante fenomeno piuttosto diffuso e in crescita, stando alle stime più recenti che parlano di 400.000 lavoratori in Italia coinvolti nello sfruttamento. È indubbio, quindi, che il legislatore debba trovare una soluzione per questi fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È una piaga sociale che talvolta rimane nascosta, soprattutto tra le campagne del nostro territorio. Uomini e donne costretti a lavorare in condizioni a dir poco non favorevoli, undici o dodici ore al giorno, spesso neanche regolarizzati, altre volte invece regolarizzati solo parzialmente, in spregio al rispetto della dignità delle persone e dei lavoratori. È giusto, ed è da me condiviso, dunque, l'obiettivo del Governo di porre fine a queste situazioni ormai inaccettabili, ma quel che non condivido è la volontà di introdurre un sistema fortemente repressivo. Mi spiego meglio: all'articolo 1 si legge che costituisce indice di sfruttamento, per cui è prevista la reclusione da uno a sei anni, anche la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro. Questa fattispecie, a mio parere, è assolutamente contraria alla *ratio* sottesa, ovvero quella di reprimere il caporalato, perché di certo non si possono includere circostanze che nulla hanno a che fare con il fenomeno, con una situazione che configura lo sfruttamento perché appare oggettivamente di minore entità. Forza Italia ha presentato alcuni emendamenti che saranno, da qui a breve, e che, se approvati dal Governo, daranno un importante contributo a una legge estremamente urgente per contrastare un fenomeno così grave e dilagante. In conclusione, quindi, ferma restando l'assoluta condivisione della necessità di contrastare il fenomeno del caporalato, va però evitato il rischio di ritenere tutti gli imprenditori agricoli responsabili di comportamenti illeciti, per evitare di penalizzare oltre misura un settore trainante per l'economia del nostro Paese.

discussione di un provvedimento che parla di caporalato e cioè di vita delle persone, di morti e di nuove schiavitù. Credo che mai come in questo caso i parlamentari debbano avere una tensione emotiva, istituzionale e di passione, qualcuno lo diceva,

vista emotivo su questi temi e noi siamo qui per risolvere queste problematiche e contrastare il fenomeno della nuova schiavitù, perché di questo parliamo.

che contiene norme positive, perché noi abbiamo bisogno di questo, cioè di promozione, come il rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che era già contenuto nella nostra normativa.

che rafforzi il collocamento pubblico e privato, al fine di garantire alle imprese agricole il reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta, perché questa è la specificità di questo tema. In un momento in cui noi stiamo realizzando una rete di politiche attive sostanziose, come quella prevista dal *jobs act*, noi abbiamo bisogno di un sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che comprenda anche i lavoratori agricoli (come è già previsto dal decreto di attuazione del *jobs act* che contenga, come ricordava la relatrice, i nominativi dei lavoratori agricoli suddivisi per territori, con dati anagrafici, contratti, inquadramento di profilo professionale. Quanto più rendiamo

per raggiungere l'obiettivo che tante più aziende possano aderire alla Rete. Si è parlato tanto di controlli. Nella Rete c'è l'Ispettorato del lavoro. Ricordiamo che l'Agenzia per l'ispettorato del lavoro riunisce più soggetti; qualcuno faceva giustamente questa opposizione, perché i controlli sono tanti e di soggetti diversi. Anche in questo caso abbiamo bisogno di

L'ultima questione che mi preme sottolineare riguarda la storia delle paghe di piazza. La collega Fabbri ricordava alcune indagini che la Commissione sugli infortuni sul lavoro del Senato ha condotto; abbiamo molto ragionato su questo fenomeno, che è molto complicato.

dovrà essere demandato alle parti sociali - una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire, in maniera adeguata, anche i fattori esterni imprevedibili che spesso condizionano l'attività del mondo agricolo. Penso che, fatta la legge, non abbiamo risolto il problema. Credo che dovremo fare in modo di avere degli alleati nella società e nel mondo della rappresentanza civile; abbiamo bisogno che la società metta in moto gli anticorpi per contrastare questo fenomeno.

come si ricordava da parte di molti colleghi, vi sono organizzazioni criminali che non scherzano, che tengono sotto ricatto intere comunità, enti locali e paesi, quindi non

Abbiamo un'esperienza, in altre zone del Paese, di automazione, di meccanizzazione della raccolta. Forse bisogna accettare la sfida a questo livello con una campagna di aggiornamento e ammodernamento del sistema.

che va dalla raccolta alla vendita, non ci sia un modo per chiamare alla responsabilità anche le imprese commerciali, le grandi distribuzioni, chiedendo loro di fare una sorta di *due diligence*? A questo proposito, onorevole Ministro, ricordo che in Commissione abbiamo approvato un ordine del giorno, che porta la firma della nostra Vice Presidente del Senato, che va proprio in questa perché noi subiamo, a volte, o comunque accettiamo l'idea di un ricatto sui costi. Ecco, secondo me, c'è bisogno di una meccanizzazione adeguata, di una *due diligence* accurata conferma delle nostre tradizioni di popolo civile, con una legislazione del lavoro. Continuo a dire che il diritto del lavoro è costituzionalizzato nel nostro Paese. Paese. È uno dei fondamenti su cui abbiamo organizzato la nostra società, e questo ci chiama a un impegno straordinario. Forse oggi abbiamo cominciato a fare un passo; non penso che abbiamo risolto tutto,

la Commissione lavoro e la Commissione giustizia. Ringrazio tutti i Gruppi che hanno contribuito in maniera propositiva e attiva a sviluppare questo disegno di legge che, a mio giudizio, costituisce un passo decisivo nella lotta al contrasto di fenomeni quali quelli che, in particolare un anno fa, vedemmo in alcune campagne del nostro Paese, che non sono certo figli di una contingenza, ma affondano radici nella storia della vicenda agricola italiana, in particolare di alcuni territori. Con le innovazioni che proponiamo

che innovare alcune strumentazioni dal punto di vista giuridico non è stato e non è affatto semplice. Giustamente è stato richiamato in questa Assemblea il dibattito che abbiamo avuto a proposito dell'articolo 603-*bis* e di come riarticolare il profilo del reato in ragione dei limiti che quell'articolo del codice penale ci ha dimostrato fin qui, della sua incapacità incapacità di rispondere alle necessità che si sono manifestate in questi anni quando si è trattato di cercare di colpire il caporalato, non riuscendoci proprio per la difficoltà di esercitare quel diritto. Considero la discussione che abbiamo sviluppato

Credo che il fatto assolutamente nuovo di specificare il reato, oltre la violenza, costituisca una novità importantissima. Ritengo altresì che l'introduzione della responsabilità del datore di lavoro sia un fatto enorme. Altro che, come abbiamo sentito anche in qualche intervento, un atto scontato di *routine* burocratico-amministrativa. Credo che l'estensione, - meglio - l'introduzione del controllo giudiziario sulle aziende con un modello che preveda la figura commissariale sia un punto di novità tutt'altro che banale e, peraltro, raccoglie una serie di spunti che ci sono stati sottoposti anche da chi lavora tutti i giorni sul versante della giustizia e coglie più di noi, probabilmente, alcune necessità. Credo che il lavoro fatto per la semplificazione degli indici di sfruttamento del reato sia, anche da questo punto di vista, una dimostrazione che la legge affonda il colpo rispetto a un'impalcatura e a una strumentazione che talvolta è rimasta sulla carta e che, quasi mai, è riuscita ad essere fino in fondo esigibile

Il settore - dal Ministero alle Commissioni - ha cercato, grazie anche alla vostra collaborazione, di guidare questa discussione. Per me questo è un fatto rilevantissimo, perché fino a un po' di tempo fa si pensava che quando si discuteva di caporalato e illegalità, in particolare nel settore agricolo, quest'ultimo si dovesse difendere da questa accusa e non dovesse invece interpretare fino in fondo la sfida di un cambiamento necessario, proprio perché la stragrande maggioranza dell'esperienza agricola italiana è fatta da imprese che, nella legalità, scommettono sulla legalità come elemento di competitività, distintività e fondante dell'impresa agricola. Penso che questa sfida vada rilanciata. Non subiamo questa grande questione, ma la vogliamo risolvere perché è anzitutto tutela

Credo anche che gli elementi nuovi presenti nel provvedimento, che si aggiungono al lavoro fatto e che richiamavo prima, siano tutt'altro che banali, anche dal punto di vista del contrasto. Quando profiliamo l'arresto in flagranza o estendiamo l'utilizzo della confisca obbligatoria, oppure quando ci poniamo il tema della responsabilità degli enti enti o definiamo la possibilità dell'assegnazione dei proventi della confisca al Fondo per le misure antitratta, noi stiamo innovando una strumentazione e lo facciamo con il massimo della possibilità che ci è data. Quindi, innoviamo in maniera significativa, così come è vero quello che è stato detto dalla relatrice, senatrice Gatti, e anche in altri interventi - con il provvedimento in esame apriamo una scommessa nuova anche nell'utilizzo di uno strumento, come la Rete del lavoro agricolo di qualità, che abbiamo impiantato con il decreto-legge n. 91 del 2014 ma che, a oggi, non abbiamo ancora verificato nel suo potenziale. Ci troviamo nel bel mezzo di una sperimentazione complicata,

di radicamento territoriale della Rete, l'unico modo che penso possa funzionare per rendere esigibile questo strumento che non può rimanere solo legato all'ambito delle attività nazionali. Benissimo che si sia fatto un lavoro per prevedere la possibilità di un ingaggio degli enti locali, in particolare su alcuni fronti. Sono stati richiamati anche prima, ma quando noi discutiamo di trasporto dei lavoratori in alcuni settori e in alcuni territori tocchiamo, come sappiamo, un nodo delicatissimo di questa vicenda. Il fatto di poter prevedere la possibilità per gli enti locali di lavorare su questo fronte, agganciandosi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, per me è un'innovazione importantissima. Benissimo aver chiarito l'aspetto delle sanzioni amministrative. Benissimo avere inserito il requisito del rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali, e benissimo, ovviamente, aver profilato l'allargamento dei partecipanti alla Rete, con tutto quello che potenzialmente può accadere in territori virtuosi, ai quali noi dovremmo lanciare una scommessa perché investano seriamente su questo strumento per provare a dare una mano a compiere il salto di qualità nel contrasto. Colgo questa occasione per richiamare il lavoro svolto parallelamente al lavoro parlamentare su questo provvedimento. Come è stato detto benissimo prima, noi non abbiamo solo aspettato il prosieguo naturale e necessario del dibattito parlamentare su questa legge per "aggredire" il nodo. siano aumentati i controlli del 60 per cento tra il 2014 e il 2015 vorrei non fosse derubricato a fatto scontato, perché anche questo dato scontato non è, figlio di una precisa volontà politica e istituzionale del Governo, del Ministero del lavoro, del Ministero della giustizia e del nostro Ministero, grazie anche alle diverse occasioni che abbiamo avuto, in Commissione e in Aula, per segnalare il tema. Per me è un fatto importantissimo avere istituito le *task force* operative su alcuni territori su alcuni territori prioritari, anche differenziando tra realtà e realtà e concentrandoci su alcune province, con il lavoro che si sta sviluppando in particolare grazie alle Forze dell'ordine, all'Arma dei carabinieri, al Corpo forestale dello Stato e agli ispettori. Per me non è un fatto banale e io sono convinto che queste *task force*, come si sta già dimostrando, stiano radicando meglio la nostra capacità di intervento, in particolare in alcune aree. Penso poi al protocollo di lavoro costituito, attraverso il Ministero dell'interno, con il Ministero del lavoro, con le Regioni e il terzo settore per la gestione sperimentale dell'accoglienza dei lavoratori stagionali, per l'assistenza in materia sanitaria, per la loro formazione e inclusione. Non cambierà tutto subito e sono consapevole che sia una battaglia di medio periodo, ma abbiamo insediato delle sperimentazioni. Io le voglio rivendicare perché sono davvero il frutto di un lavoro comune. Non si risolverà tutto con questa legge: è vero. il nostro ruolo, il nostro lavoro e il nostro compito è quello di fare buone leggi e, dal Parlamento e dal Governo, contribuire a sviluppare sempre di più una strumentazione all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte, nella consapevolezza che stiamo parlando di un grandissimo tema che, a mio giudizio, va ben oltre il settore. il settore. Se l'esperienza agricola riesce a innovarsi sul piano della legalità, del lavoro buono, sperimentando strumenti che certificano quanto in realtà buon lavoro e esperienza agricola siano uniti, noi facciamo un mestiere utile non solo per i lavoratori più coinvolti e per le imprese agricole più coinvolte (questo, prima di tutto), ma segniamo, in maniera assolutamente positiva, un'esperienza nazionale e contribuiamo a sviluppare, secondo me al meglio, anche la responsabilità che ci compete. È vero

2382** Presidente, onorevoli colleghi,

ossia che viaggiando in mare su barconi fatiscenti e gremiti all'inverosimile, in mano a spregiudicati scafisti senza scrupoli, si corre il rischio della vita. davvero di una grande scoperta questa del Ministro, veramente degna di un illuminato *leader* politico. Possibile che nessuno ci avesse pensato prima?

in grado di dare risposte alle esigenze dei tanti amministratori locali che sono purtroppo destinatari di questa politica inefficace e che, soprattutto in alcuni piccoli centri, devono fronteggiare un'emergenza che lo Stato, fino ad oggi incapace di trovare soluzioni, scarica sul territorio. Ho avuto modo di sentire il ministro Alfano l'altro giorno su «Radio anch'io», trasmissione

hanno uno stile di vita diverso. Permettetemi: non paragoniamo gli emigranti italiani con questi migranti solo per un fatto di dignità e non per discriminazione. Se questo è il concetto che il Ministro ha dei nostri italiani e dei migranti, ahimè, è bene che cambi mestiere.

la nostra mozione di revoca del cavalierato a Mauro Moretti, all'epoca dei fatti amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Scrissi anche una lettera aperta a tutti senatori toscani, di tutte le forze politiche, sicura che non sarebbe mancata la condivisone e la sottoscrizione della mia mozione finestra"), presentata già nel 2014, per rispetto del dolore dei familiari della strage di Viareggio e di tutti i morti sul lavoro del personale delle Ferrovie. Successivamente, sulla base della mia richiesta di revoca, alla Regione Toscana, grazie ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, quest'anno è stata approvata una mozione all'unanimità, per chiedere allo Stato di fare altrettanto. Intanto diciamo che è molto grave e mi duole denunciare che a oggi nessuna firma al Senato è stata aggiunta da nessun nuovo senatore, di di nessun altro partito. Nessuno più ha apposto la sua firma a una richiesta più che legittima, che non si basa esclusivamente sulle vittime della strage di Viareggio, per la quale Moretti è imputato - con profonda tristezza ricordo che il cavalierato fu riconosciuto da Napolitano a soli undici mesi dalla strage di Viareggio - ma soprattutto per la follia di aver aver riconosciuto cavaliere del lavoro colui che dietro di sé si era lasciato una scia di morti e feriti inaccettabile: nella nostra mozione l'elenco è ben dettagliato. La gestione di Moretti fu tutt'altro che positiva per i lavoratori: per sistemare i bilanci in passivo del gruppo Ferrovie dello Stato, fece tagli pesanti sul personale e sulla manutenzione, non investì sufficientemente in prevenzione e sicurezza sul lavoro. Le conseguenze furono pagate da semplici cittadini, da passeggeri e dai lavoratori delle Ferrovie (macchinisti, operai, addetti alla manutenzione, eccetera). Più di 100 sono state le vittime durante la sua gestione, spesso spesso causate da gravi carenze e mancati investimenti nella sicurezza ferroviaria. Quindi, ci chiediamo quali siano stati i meriti per premiarlo e definirlo cavaliere del lavoro. che come senatrice e cittadina non condivido chi fa orecchie da mercante e alle commemorazioni si riempie di cordoglio, ma poi nei fatti non muove un dito. La politica deve dare un segnale forte e non solo fare annunci e preghiere, signora Presidente. Altrimenti, coloro che chiedono di vivere in un Paese normale verranno beffati due volte. Senatori, come potrete presentarvi davanti alle associazioni dei familiari delle vittime, di tutte le vittime di Ferrovie dello Stato, se non avete il coraggio delle vostre azioni? Nel processo per la strage di Viareggio, oltretutto, pende una spada di Damocle: la prescrizione. Che almeno qualcuno, qualcuno, pubblicamente, suggerisca a Moretti di non avvalersi della prescrizione. Chiediamo un atto politico forte, affinché sia fatta piena giustizia, qualunque essa sia. A questo punto, noi del Movimento 5 Stelle scriveremo una lettera aperta al presidente Mattarella e al ministro dello sviluppo economico speranza che questa richiesta possa essere accettata. Mai vorremmo pensare che in questo Paese ci sia l'ordine del sacrificabili e quello degli intoccabili. Esorto i familiari delle vittime a contattare uno ad uno i senatori che non hanno aderito alla nostra pubblica richiesta e a farsi dire le motivazioni della loro ritrosia a

oggi, 28 luglio, è la giornata mondiale contro l'epatite C. Anche se in un'Aula purtroppo quasi vuota, credo che ricordare questa data possa dare un piccolissimo contributo, per fare in modo che ci sia un po' più di attenzione rispetto ad alcune patologie, che sono importanti e che stanno creando una grande preoccupazione e rischiano di diventare un tema drammatico, non soltanto per il nostro Paese, ma anche per molti altri Paesi, pur ricchi e facenti parte del mondo sviluppato. Da pochissimi anni abbiamo dei farmaci, che sono estremamente efficaci per questa patologia - la loro efficacia è sicuramente superiore al 90 per cento dei casi trattati che sono immessi in commercio a prezzi altissimi. Ciò fa sì che si ponga, per la prima volta in Paesi come l'Italia, il problema di come garantire l'accesso a questi farmaci per tutti i cittadini che potrebbero trarne vantaggio. Ricordo soltanto che in Italia c'è oltre oltre un milione di malati, portatori cronici del virus dell'epatite C, e di questi circa 330.000 hanno la cirrosi.

sacrificare troppo tempo dell'Assemblea a questo argomento e per sottolineare l'importanza del problema, osservo che il Senato degli Stati Uniti d'America ha svolto un'inchiesta su questo tema, perché il problema è molto grave anche per Paesi ricchi come gli Stati Uniti, e ha e ha concluso, perlomeno con riguardo al primo farmaco che è stato immesso in commercio da una multinazionale, che il costo così elevato del farmaco

il prezzo così alto è legato semplicemente alla ricerca del massimo profitto da parte dell'azienda, che si comporta più come un'azienda finanziaria speculativa che non come un'azienda che produce farmaci che possono salvare una vita umana. Di fronte a queste affermazioni, che ormai stanno diventando di dominio comune nella letteratura specialista ma anche nel mondo della comunicazione, l'Italia deve essere in grado di affrontare questo tema in modo adeguato. L'AIFA ha negoziato il prezzo del farmaco alla fine del 2014, un prezzo che è molto elevato e che sappiamo essere ancora secretato. Il contratto è già scaduto, però l'AIFA dichiara di non essere in grado di portare rapidamente a compimento una nuova

L'abbiamo scritto l'anno scorso nella legge di stabilità, all'articolo 1, comma 570; a questo comma non è ancora stata data attuazione (abbiamo recentemente chiesto indicazioni). Ci troviamo di fronte a pazienti che, per poter essere trattati, devono diventare gravi e solo quando sono gravi possono essere trattati. Un Paese civile non se lo può più permettere e io credo che di queste cose dobbiamo essere assolutamente consapevoli. al Presidente e all'Assemblea del Senato un accorato appello, affinché questo diventi argomento sul quale si ponga l'attenzione di tutti i decisori e della popolazione, affinché lo si possa affrontare, anche perché è il banco di prova di è il banco di prova di cosa succederà quando, fra breve, entreranno in commercio decine di farmaci antitumorali ad altissimo costo, rispetto ai quali non potremo improvvisare la risposta.

finestra"), inerente a una sentenza recentissima (17 giugno scorso) del TAR della Lombardia. Cosa ha fatto il TAR della Lombardia? Ha dato ragione alle società che estraggono in Italia, in questo caso gas. Queste società molto semplicemente hanno detto: «Cara Italia, vi stiamo pagando troppe *royalty*, vi stiamo pagando il 20 per rispetto a quelle che secondo noi erano dovute negli ultimi due anni». Hanno fatto tutto un ragionamento tecnico e alla fine il TAR gli ha dato ragione. Ora, se il MISE o il MEF non ricorrono in Consiglio di Stato, Comuni e otto Regioni dovranno restituire il 20 per cento delle *royalty* incassate negli ultimi due anni. Noi già abbiamo un regime di *royalty* che esenta le compagnie dal pagare fino a una certa franchigia grazie a questo, metà dei pozzi non pagano nulla, perché sono così intelligenti da rimanere sotto la franchigia. Già siamo in regime di esenzione per le produzioni ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca. Quindi basta che io prolunghi questo regime e continui a estrarre; con la scusa che sono in regime di prova, non pago assolutamente nulla. A me verrebbe da dire: della serie «cornuti e mazziati».

tra il gas e gli altri idrocarburi. Se manca questa distinzione non siamo in grado di verificare quali sono le *royalty* del solo gas, e non siamo neanche in grado di avere un minimo di trasparenza. Inoltre, sono indicate le estrazioni lorde, non quelle nette.

La seduta è tolta